la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha organizzato i tempi del dibattito sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'emendamento interamente sostitutivo del disegno di legge di conversione del decreto-legge sulla manovra economica. Per la discussione generale sulla fiducia, che si esaurirà nella seduta pomeridiana odierna fino alle ore 21,30, sono state assegnate ai Gruppi 5 ore e 15 minuti, così ripartite: PdL 30 minuti; PD 2 ore e 30 minuti; Lega Nord 30 minuti; IdV 40 minuti; UDC-SVP-Aut (UV-MAIE-IS-MRE) 30 minuti; Misto 30 minuti. Le dichiarazioni di voto avranno luogo domani mattina alle ore 9,30. Pertanto, la chiama dei senatori avrà inizio intorno alle ore 10,30. Seguirà, sempre nella seduta antimeridiana di domani, 1'esame del decreto-legge in materia ambientale, approvato dalla Camera dei deputati. Qualora la discussione del provvedimento dovesse concludersi entro le ore 14 di domani, la seduta pomeridiana non avrà luogo. In tal caso la commemorazione di Rina Gagliardi si svolgerà in apertura della seduta pomeridiana di martedì 20 luglio. È stata altresì sconvocata la seduta antimeridiana di venerdì 16 luglio. Si ricorda che domani, alle ore 14,30, è convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di otto componenti del Consiglio superiore della magistratura. La Conferenza dei Capigruppo ha inoltre definito il calendario dei lavori per la prossima settimana che prevede, a partire dalla seduta pomeridiana di martedì 20 luglio, i seguenti argomenti, oltre all'eventuale seguito del decreto-legge in materia ambientale: decreto-legge sulla regolarità del trasporto marittimo; documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari; decreto-legge recante misure urgenti in materia di energia; disegno di legge sulla riforma universitaria. Per i decreti-legge in calendario i tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi. La definizione del prosieguo dell'*iter* del disegno di legge sulla riforma universitaria sarà stabilita dalla prossima Conferenza dei Capigruppo. Nel corso della prossima settimana sarà inoltre ricordata la figura di Egidio Sterpa. Infine, è stata rappresentata al Governo la richiesta della Presidente del Gruppo del Partito Democratico di prevedere un dibattito, con la presenza del Presidente del Consiglio dei ministri, sulle vicende connesse alla cosiddetta inchiesta sull'eolico.

nella seduta antimeridiana il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento 1.10000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge al nostro esame

formali, voglio riferire, signora Presidente, esattamente sugli esiti della Commissione. Due sono state le questioni poste. Per un verso, l'apprezzata ed unanime coincidenza con il patto politico che era stato stretto in Commissione, visto che l'emendamento del Governo non ha affrontato

non grande rilievo).

La norma è stata riproposta in modo identico in questo emendamento, né alla stessa è stata associata un'altra copertura: il Governo, cioè, ha sostanzialmente ritenuto di dover riproporre la norma, e senza copertura. Per quel che mi riguarda posso solo osservare che, in effetti, il dibattito in Commissione andò esattamente nei termini

l'utilizzo del Fondo unico di giustizia non ha costituito sul piano del merito occasione di giudizio. Probabilmente è apprezzabile da parte di tutti, ma i colleghi

che hanno riguardato altri punti del testo elaborato in Commissione, e sotto questo profilo sono in effetti più efficaci.

di esaminare la questione che è stata posta dal Presidente della Commissione bilancio, esattamente nei termini in cui il Presidente della Commissione bilancio l'ha formulata. Noi siamo in presenza, signora Presidente, di un comma inserito nel testo al nostro esame, precisamente all'articolo 6,

di un emendamento del relatore presentato a questo scopo, allorché la Commissione bilancio decise unanimemente di non procedere all'approvazione dell'emendamento in questione appunto che esso determinasse problemi seri di corretta copertura finanziaria. signora Presidente. Stiamo parlando dell'articolo 6, comma 21-*quinquies*, che è esattamente l'oggetto della relazione fatta poco fa dal presidente Azzollini. In epoche diverse, con Presidenti diversi, in presenza di relazioni di questo tipo del Presidente della Commissione bilancio, la Presidenza ha disposto, d'accordo col Governo, l'espunzione della parte di maxiemendamento in questione dal testo su cui avviare la discussione. Voglio insistere perché si tratta di questione assai seria. Cosa dice questa norma? Altrimenti sembra che parliamo di cose formali che non hanno fondamento. Dice esattamente che

alienazione effettuata sul mercato debbono essere riversati immediatamente sul Fondo unico giustizia, che è un Fondo che finanzia direttamente le spese di giustizia.

i proventi della vendita vengono messi nel Fondo unico giustizia. Nel momento in cui stanno là, quei proventi danno luogo immediatamente a spesa, ma i titoli sequestrati possono essere, così come sono stati sequestrati, oggetto di dissequestro. Dal punto di vista della loro classificazione, come dobbiamo considerare quei proventi che derivano dalla vendita del titolo sequestrato in prima istanza? Li dobbiamo classificare come debito. La domanda che si pone è molto semplice: si può un'innovazione legislativa aumentando il debito sul debito? Naturalmente la risposta è no, e, a mio giudizio, si pone un serio problema di rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione a proposito di questa norma,

Presidente, di questo tema si è già parlato in Commissione, e già il Governo aveva ipotizzato e presentato

la capienza di questi Fondi è particolarmente ampia, così ampia che l'eventuale importo che dovesse essere retrocesso

Presidente, io non sollevo nessun problema riguardo a nessun rischio. Le leggo, così almeno è chiaro, cosa ha scritto il Servizio del bilancio, e non Enrico Morando, bieco oppositore, a proposito di questo comma: «Al riguardo, andrebbe valutato un eventuale impatto sui saldi di finanza pubblica legato alle incertezze circa il trattamento contabile delle entrate rivenienti dall'alienazione in discorso secondo le regole di SEC95. Tenuto conto, infatti, dell'incerta titolarità giuridica dei cespiti in questione, qualora tali entrate non potessero essere imputate al conto economico della PA o lo fossero con un disallineamento temporale verrebbero registrate solo le uscite legate all'utilizzo dei proventi con conseguente aggravio dell'indebitamento». Non è un'opinione, è un fatto: questo comma così com'è non può stare in un provvedimento che voglia rispettare l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Senatore Morando, capisco perfettamente, però il Presidente della Commissione bilancio non ha fatto nessuna proposta di espungere alcunchè.

il Presidente della Commissione bilancio ha appena riferito che questo identico testo è stato presentato come emendamento alla Commissione bilancio e che questa unanimemente lo ha dichiarato

dal senatore Morando. Il Governo ha comunicato al Presidente del Senato che, alla luce della relazione del presidente Azzollini sui lavori odierni della Commissione e pur prendendo atto delle osservazioni avanzate in Aula

questa occasione. Ricordo che il presidente Pera e il presidente Marini hanno sempre rispettato questo principio. Il presidente Schifani lo vìola: evidentemente avrà valutato che per il decoro del Senato è meglio così. quello che abbiamo avuto di fronte in questo mese di confronto in Commissione bilancio è un Governo paralizzato dalla paura: paura della sua maggioranza, innanzitutto. Il Governo ha scelto di esorcizzare questa paura premiando le spinte corporative e penalizzando le istanze di cambiamento e di riforma, che pure nella maggioranza sono assai vivaci:

Altro che sindacato del territorio, signora Presidente: in questo caso, il sindacato che viene alla memoria è piuttosto quello di Jimmy Hoffa! paura di un confronto aperto con l'opposizione. Anche in questo caso il Governo ha scelto di accogliere qualche proposta di aggiustamento ai margini delle misure di risparmio, ma si è sottratto al confronto vero su scelte vere di cambiamento. Il ripristino - udite, udite! - dei riposi compensativi dei dipendenti pubblici (generali, colonnelli e così via) per la partecipazione ai convegni, sì; la riduzione strutturale del prelievo IRPEF sulla quota di salario da contrattazione di secondo livello, quella no. Con tanti saluti agli operai di Pomigliano che rischiano del loro e hanno approvato il recente accordo! paura del Paese e delle istanze più innovative che in esso si agitano: la riforma del trattamento fiscale degli affitti pagati e percepiti per favorire la mobilità dei fattori sul territorio e combattere l'economia sommersa, no;

In quarto luogo, vi è la paura della trasparenza, anche là dove - come sulla tenuta e la gestione dei conti pubblici - essa rappresenta un bene pubblico fondamentale per un Paese che ha il terzo debito pubblico del mondo.

a disposizione di quelle intese tra Presidente della Camera e Presidente del Senato, previste dalla legge di contabilità, che possono costituire il primo passo per la costruzione anche in Italia di quell'Ufficio del bilancio del Parlamento che è indispensabile per garantire a tutti la credibilità e l'affidabilità dei nostri dati di finanza pubblica e al tempo stesso per realizzare un salto di qualità nel lavoro parlamentare, soprattutto in vista dell'attuazione della legge sul federalismo fiscale? La risposta purtroppo è sempre la stessa. Solo un Governo forte e autorevole, quale il Governo italiano sa ormai di non essere, può rinunciare al monopolio della conoscenza in nome di un bene pubblico superiore. Solo chi è forte per sé e in sé, e si sente forte, è in grado di rinunciare al monopolio della conoscenza, in nome della costruzione di un soggetto che possa dargli credibilmente torto, garantendo a tutti gli operatori, a tutti i soggetti, a tutti gli osservatori internazionali l'affidabilità e la credibilità dei conti pubblici.

la maggioranza parla solo per bocca del relatore, oppure illustra con autorevolissimi suoi esponenti emendamenti che, se approvati, disegnerebbero una manovra totalmente altra rispetto a quella del Governo; soluzioni e interventi - ho già fatto qualche esempio in proposito - che sono parte essenziale del programma del Popolo della Libertà che, proposti al voto dall'opposizione, vengono respinti con il solo argomento che non sarebbe questa la sede giusta per la loro soluzione, salvo poi concludere che questa sede è perfettamente ospitale per interventi di cui non si è mai discusso in precedenza e che non hanno alcuna influenza significativa sui caratteri e sulla dimensione della manovra. Questa paura che caratterizza il Governo compromette le *chance* del Paese, delude le sue energie migliori e per questa via affievolisce la speranza e la fiducia, i veri motori del cambiamento del Paese.

avrebbe bisogno della sua migliore politica da entrambi i lati dello schieramento per essere guidato nella difficile azione di superamento dei due pesi che ne ostacolano la corsa:

produttività dei fattori e del lavoro, in crescita stentata ininterrottamente da 15 anni. La politica dal lato del centrodestra risponde però al Paese con lo spettacolo di Ministri nominati al solo scopo di evitare di comparire in processi in cui sono imputati; con la corruzione predatoria che invade anche il segmento più nobile e popolare della nostra pubblica amministrazione, ovvero la Protezione civile; con cene con cene che - anche previo il coinvolgimento di autorità morali e di garanzia, la cui autonomia è parte essenziale del capitale di credibilità del Paese

Il Gruppo del Partito Democratico in Commissione bilancio ha prima delineato nelle sue linee essenziali, nella discussione generale, e poi tradotto in una ventina di emendamenti fondamentali - quelli che contano davvero - una linea di intervento sui problemi del Paese tanto rigorosa nell'aggiustamento dei conti quanto coraggiosa nella promozione del cambiamento necessario per rilanciare la qualità e la quantità dello sviluppo. È un altro discorso al Paese, fondato su quattro capisaldi essenziali, che qui posso solo richiamare per cenni. In primo

Se accettassimo la proposta della Germania di maggiore rigore fiscale sui singoli Stati nazionali, fino al limite dell'introduzione in Costituzione o tramite il Patto di stabilità di vincoli numerici al *deficit* in rapporto al prodotto,

per quella di gestione del debito pubblico di tipo europeo, il sistema europeo si troverebbe ad affrontare la competizione globale come il pugile che affronta l'incontro valido per il titolo mondiale facendosi legare una mano dietro la schiena. Sarebbe inaccettabile, ed è incredibile e malinconico dover constatare che una grande Nazione come la Germania è oggi diretta da un Governo e da un *premier* che non ha la generosità e la visione dei grandi Kohl, dei grandi Schröder, che hanno saputo cambiare quel Paese in nome dell'europeismo. luogo, la corsa sfrenata della spesa corrente primaria della pubblica amministrazione va assolutamente fermata: subito, costi quel che costi. Essa, infatti, è all'origine sia dei problemi di efficienza del Paese (spendiamo come e più di altri per assicurarci prestazioni essenziali al buon funzionamento dell'economia, come giustizia, sicurezza, ordine pubblico, ma otteniamo molto meno degli altri) sia degli abissi di disuguaglianza che lo caratterizzano. In Italia, con una spesa sociale attorno al 25 per cento del prodotto, noi riusciamo a ridurre la vulnerabilità sociale solo del 53 in Francia, con una spesa sociale di due soli punti superiori, la vulnerabilità sociale viene abbattuta del 70 per cento: 17 punti in più! Ora, noi abbiamo dimostrato che c'è un altro modo rispetto a quello scelto dal Governo per abbattere la spesa corrente: uscire dal ristretto ambito della spesa rimodulabile, aggredire il 100 per cento della spesa con revisione sistematica, valutazione dei risultati, definizione di precisi obiettivi di medio-lungo periodo su basi comparative, responsabilizzazione dei dirigenti politici e amministrativi, premi per chi merita e durissime penalizzazioni per chi non è capace di fare il suo mestiere. Senza guardare in faccia nessuno, prefetti o non prefetti, e senza accettare ricatti da nessuno. bisogna restituire ai contribuenti leali almeno metà del gettito riveniente dalla lotta all'evasione fiscale, scegliendo tra i contribuenti secondo il punto di vista di chi vuole al tempo stesso più efficienza, più libertà e più eguaglianza. Giù le aliquote IRPEF sui redditi da lavoro delle donne, e giù di parecchio: secondo me è la migliore delle scelte possibili a questo proposito. all'apertura dei mercati chiusi per fare posto alla concorrenza e al merito, senza il quale i nostri giovani hanno un destino privo di futuro e di dignità, l'alleviamento del peso soffocante della burocrazia sotto il quale perisce nella competizione internazionale una parte importante delle nostre imprese. abbiamo sfidato il Governo e la maggioranza a fare finalmente sul serio, a puntare al bersaglio grosso, a cercare di agguantare una volta tanto l'arrosto, non accontentandosi del profumo. separazione proprietaria immediata di Rete Gas da ENI e all'autocertificazione garantita da agenzie private per i rapporti fra imprese piccole e medie e pubblica amministrazione. Il Governo e la maggioranza ci hanno proposto un importante dibattito sull'articolo 41 della Costituzione. Campa cavallo! Questa è la politica di bilancio ed economica che il Partito Democratico ha proposto nel corso di questo dibattito, come dimostrano gli emendamenti che abbiamo presentato, e di cui tutti si possono rendere conto. Altro che muro di no e rifiuto del rigore fiscale di cui parla il Presidente del Consiglio! Distorcere il senso delle proposte dell'avversario è sempre - sempre - segno di debolezza, e il Presidente del Consiglio oggi, purtroppo per il Paese, è molto debole. Noi abbiamo detto che una manovra è necessaria, che la correzione netta di 25 miliardi - 15 da minori spese e 10 da maggiori entrate - è sostanzialmente corretta. Abbiamo però aggiunto che essa è gravemente insufficiente per il rilancio delle nostre capacità competitive e per garantire un adeguato livello di coesione sociale in un Paese che, tra quelli dell'OCSE - 30 Paesi, tra cui Turchia e Messico, per

dal Messico, dalla Turchia e dagli Stati Uniti d'America. Poi veniamo noi, un grande Paese che sta nell'Europa, dove c'è il modello sociale europeo. Per livelli di disuguaglianza siamo *recordmen* non solo in Europa, ma tendenzialmente tra i Paesi sviluppati nel mondo. Per questo, abbiamo proposto di portare la manovra lorda a 30 miliardi, con altri 5 miliardi di risparmi realizzati secondo quel metodo di intervento che ho prima descritto. Abbiamo poi proposto di usare i 5 miliardi rivenienti da questa operazione per ridurre, esattamente della stessa cifra, la pressione fiscale sui contribuenti leali. inoltre avanzato la proposta della riduzione dell'IRPEF sul reddito da lavoro delle donne, che ha come alternativa praticabile, se la maggioranza avesse scelto questa strada,

Chiede fiducia per sé, ma così facendo, purtroppo, toglie fiducia in se stesso al Paese. Noi voteremo no.

(lasciamo stare etiche) politiche del Paese, perché è una risposta al senso profondo della coesione nazionale, ad una delle ragioni dello stare assieme, della configurazione del nostro Stato democratico. Avendo ascoltato il senatore Morando e ricordando le parole del relatore di minoranza, debbo dire ai rappresentanti del Governo che

dall'inizio della legislatura, in particolare dopo l'esplosione della crisi finanziaria. È stato ora ribadito che,

Ritengo che un Ministro del tesoro, come mi piace chiamarlo, faccia bene a preoccuparsi di queste cose. La cosa impensabile per un Paese nelle condizioni dell'Italia è quella di non accompagnare una simile politica con uno sforzo di tenuta, in particolare della domanda interna. Lascio stare le condizioni per lo sviluppo, per la ripresa, per una maggiore competitività del Paese, che vede arretrare le retribuzioni in tutti i settori: noi non siamo cresciuti al livello degli altri Paesi europei per questa stagnazione della domanda interna, perché fin quando il mercato internazionale ha tirato, uno dei punti di forza del nostro Paese è stata la capacità della piccola e media impresa di tenere i mercati esteri.

Alla fine, sia pure con uno stanziamento molto limitato (45 milioni di euro), passò l'idea di una zona franca che aveva precedenti storici in altri terremoti che potesse contribuire alla ricostruzione e al riavvio dell'area delle piccole imprese che hanno costituito uno dei punti fondamentali del bilancio della città dell'Aquila.

90 milioni di euro sono una cifra che potrà consentire, almeno lo spero, con il riavvio della ricostruzione della città dalla fine di quest'anno e certamente e necessariamente dall'anno prossimo, con uno sforzo di programmazione che deve recuperare i ritardi che vi sono stati,

ma in 120 mensilità. Resta il fatto che quanto ha prodotto una calamità nazionale così grave e dolorosa

la possibilità di riaprire una città, un mondo che non si può sottrarre alla ricchezza dell'Italia, credo che dovrebbe essere quasi la normalità

onorevoli colleghi, dopo una serie infinita di dichiarazioni da parte di questo Governo, sulla base delle quali si è ripetutamente premurato di dirci che la crisi economica era ormai alle spalle, e dopo aver tacciato di pessimismo (peggio, catastrofismo) ogni voce che aveva timidamente tentato di dissentire da una così rosea visione, ci troviamo nuovamente ad affrontare con l'ennesimo voto di fiducia una manovra finanziaria che prevede tagli per un ammontare di circa 25 miliardi di euro. Si tratta decisamente di una cifra non da poco per un Paese che si trova con la crisi alle spalle. Questa manovra colpisce esclusivamente la parte più debole del tessuto produttivo del Paese. Pertanto, all'indomani saremo inevitabilmente ancora più poveri e più deboli, senza un chiaro indirizzo di sviluppo industriale, con un tessuto produttivo ridimensionato, con un mercato del lavoro privo di adeguati strumenti di riqualificazione e sostegno. Non affrontate nessuna delle emergenze che ci attanagliano: la caduta della ricchezza nazionale, la crescita della disoccupazione, le difficoltà del tessuto imprenditoriale e la perdita di potere d'acquisto dei redditi di lavoro e di pensione. Di sviluppo non ve ne occupate neanche a parlarne, o meglio ve ne occupate per mortificarlo con norme, come quella sui certificati verdi, che bloccano gli investimenti già impostati con un danno gravissimo sul piano dell'innovazione e del miglioramento della bilancia energetica del Paese; una misura che avrà inevitabili ripercussioni sullo sviluppo delle imprese del settore interessate a progetti (biomasse e biogas, eolici, geotetermici ed idroelettrici), pregiudicando così la tenuta di una delle poche filiere in crescita che il nostro Paese vanta e con inevitabili ricadute occupazionali. Venendo più specificamente al settore dell'agricoltura, di cui mi occupo, avete previsto un taglio di spesa di ben 58,2 milioni di euro, due terzi dei quali riguardano gli investimenti. Voglio ricordare all'Assemblea che, se a queste riduzioni si sommano i tagli già operati in questi due anni di legislatura dalle scorse finanziarie, c'è da chiedersi per quale scopo mantenere in vita questo Ministero che avete completamente svuotato di significato. La totale mancanza di misure di indirizzo e sostegno al settore, diversamente da quanto fatto dai principali Paesi europei - Francia, Spagna e Germania in testa - che considerano, diversamente da voi, il comparto agricolo come una risorsa da tutelare e sulla quale investire, dimostra ancora una volta, nel caso ve ne fosse bisogno, la completa assenza di una progettualità a medio-lungo periodo, quale dovrebbe invece caratterizzare una manovra strategica per lo sviluppo. Non vi curate di questo settore, e lo fate anche con una norma abbastanza superficiale promettendo, con balletti esasperanti, misure che già sapete di non prevedere. Penso all'interminabile vicenda del rifinanziamento del settore bieticolo-saccarifero, rimandando, con un crudele balletto, di provvedimento in provvedimento le speranze di sopravvivenza dei lavoratori di questo comparto. Mandate al macero migliaia di operatori non prorogando le agevolazioni contributive agricole delle aree svantaggiate di montagna in scadenza il prossimo 31 luglio.

soprattutto alle coltivazioni sotto serra. Per non parlare poi della predisposizione dei decreti attuativi dell'*Authority* nazionale sulla sicurezza alimentare. Lo voglio ricordare ai colleghi qui in Aula: ci siamo scandalizzati per i pomodori cinesi, per la mozzarella blu, blu, ma non sappiamo che in Italia non esiste nessuno che si occupi della sicurezza alimentare degli italiani. Stiamo attendendo da due anni i decreti attuativi di questo Governo; anzi, un mese fa

e sono dovute intervenire tutte le istituzioni italiane per la sua salvaguardia. Ancora oggi siamo in attesa dei decreti attuativi. Ne ha parlato il presidente Marini poc'anzi: vede, Presidente, appartengo a una terra che ha subito un terremoto nel 2002 a cui fu riconosciuta la decontribuzione per quell'anno, da restituire in 24 anni. Ebbene, questo Governo ha onorato solo i primi sei anni, poi ci ha completamente dimenticati. Anzi, l'INPDAP lo scorso mese ha chiesto la restituzione immediata di questi contributi, e solo il Comune di Foggia deve restituire 15 milioni di euro. 15 milioni di euro. Poi abbiamo avuto il terremoto dell'Umbria, altra dimenticanza, e siamo arrivati al terremoto dell'Abruzzo. Però - e questo è il miracolo vero - il vostro Ministro dell'economia e delle finanze riesce a scovare i soldi necessari a prorogare il pagamento delle multe per le quote latte per 67 - sottolineo 67 - splafonatori, grandi elettori di un partito rappresentato in quest'Aula. Ed è lo stesso partito che ha premuto per la prima legge del 2003 (prima rateizzazione) per la seconda legge, che abbiamo votato lo scorso anno (la legge Zaia del 2009), che prevedeva la seconda rateizzazione per coloro che non avevano pagato sette anni prima. Ebbene, in questo provvedimento che cosa succede?

Voglio solo ricordare che le multe ci sono costate 2 miliardi, 1 miliardo coperto dai fondi FAS. A tale proposito avevamo presentato una serie di norme per le agevolazioni contributive, ovviamente respinte da questa maggioranza, e neanche gli appelli del ministro Galan vi hanno smosso, né tantomeno vi siete preoccupati di mandare in Europa un Ministro che avete privato della necessaria autorevolezza per affrontare l'intera partita della riforma della PAC, la politica agricola comune. Addirittura,

che vi permetterà di andare avanti di proroga in proroga. Poi scrivete - non so chi scrive, perché non sono riuscita a capire - anche di accertamenti in corso. Cosa vuol dire? Che nel 2003 e nel 2009 vi siete sbagliati? Restituirete i soldi a coloro che hanno già pagato, o sarà soltanto un provvedimento per non far pagare questi 67 signori? Questo è il dato. dato. Oggi incassate i ringraziamenti dei senatori della Lega, grati per la sensibilità mostrata nei confronti del mondo agricolo. La vostra delegazione di europarlamentari esce con una nota in cui chiede al Parlamento italiano di rispettare la legalità e di non esporre i cittadini italiani al pagamento di una nuova maximulta. Ma evidentemente tutto questo non ha avuto riscontro. Ripeto e concludo: non è un provvedimento a favore dell'agricoltura italiana non è un provvedimento, a favore degli allevatori onesti, non è un provvedimento soprattutto per un settore in crisi quale il lattiero-caseario: è un provvedimento per alcuni amici di questa maggioranza che ancora una volta non hanno fatto altro che mortificare le esigenze di un'agricoltura fortemente in crisi. E oggi, cara Presidente, gli allevatori e gli agricoltori italiani ringraziano.

intendo intervenire in questo dibattito sulla questione di fiducia posta dal Governo per molteplici ragioni. In primo luogo, per ringraziare i colleghi del Gruppo dell'Italia dei Valori, in particolar modo il senatore Mascitelli, che è stato puntualmente presente per illustrare e cercare di integrare e modificare una manovra brutta e scadente. per evidenziare che ancora una volta il Governo e questa maggioranza sono in trincea con l'elmetto per difendersi da se stessi.

Quindi, è una manovra confusa, raffazzonata, improvvisata, come illustri economisti hanno rilevato, che ha esibito grandi numeri cercando di offrire un quadro macroeconomico rassicurante, le famose lacrime e sangue: ma queste e quello sono per i pochi, sempre per i soliti. Chi paga davvero con questa manovra miope sono i giovani, colpiti dal taglio dei contratti a tempo determinato e dal blocco delle assunzioni e delle carriere nel pubblico impiego che, come noto, va a penalizzare proprio chi è entrato da poco e con salari bassi. Ovviamente, ed ancora una volta, non essendo una manovra che ha guardato strutturalmente al bilancio dello Stato, la riforma degli ammortizzatori sociali la leggiamo soltanto sulle vignette dei giornali. L'assestamento strutturale langue del tutto. È una manovra economica fondata sui refusi, anche sulle brutte figure che, per contratto stipulato con la sua maggioranza, ha fatto il relatore, che ha presentato gli emendamenti li ha commentati e li ha cancellati; poi, ancora una volta, ha cercato di illustrarli. Vedete, questa è una manovra che non risolve nessun problema e di cui nel 2012, se ci andrà bene, non rimarrà traccia.

Corte dei conti e Confindustria stimano in oltre 120 miliardi di euro il buco dell'evasione fiscale, il Governo si preoccupa di recuperarne Questo Governo, quindi, non vuole fare la lotta all'evasione fiscale. Questo è un dato politico certo, ineludibile ed incontestabile: abbiamo da che parte sta. Le uniche norme accettate sono quelle poste all'attenzione da un *supporter* del Presidente del Consiglio e di questa maggioranza, come si è manifestata la Presidente di Confindustria. Sono soltanto pochi spiccioli quelli che andiamo a recuperare all'evasione fiscale. Era questo il nocciolo, così come anche il nocciolo duro è la lotta ai fenomeni corruttivi. Ovviamente questo è un Governo parolaio, una maggioranza chiacchierona che vende fumo, se non veleni tossici: presenta un disegno di legge anticorruzione, ma ovviamente non può portarlo avanti perché al suo interno, nel Governo, nella maggioranza e nel Parlamento ci sono componenti autorevoli che in queste cose ci sguazzano, e ci guazzano in maniera devastante per la credibilità del Parlamento e, se consentite, della medesima maggioranza! Su questo pensavamo che la maggioranza avrebbe finalmente, come fa qualche persona pure colpevole, portato avanti atti di resipiscenza operosa; speravamo in una sorta di conversione sulla via di Damasco: peccare si può, ma quantomeno ci vuole un minimo di conversione al momento opportuno. Invece non abbiamo nulla, neppure misure a sostegno dell'occupazione. Abbiamo una manovra che contiene misure depressive,

- lo sappiamo e lo sapete, colleghi della maggioranza - che hanno difficoltà a sbarcare il lunario. È una manovra complessa, al di là dei giudizi che ci vengono dalle autorità europee e internazionali. Non stiamo discutendo dei saldi: nessuno dice che la manovra non andava fatta; la manovra andava fatta, la manovra andava fatta, ma con delle misure che rilanciassero la speranza di questo Paese. Invece, dopo oltre 40 giorni,

il Parlamento partorirà un topolino e alla fine l'unico risultato che sarà stato raggiunto è quello di aver quantomeno cercato di illustrare e puntualizzare gli errori; nel nostro caso presentando una manovra diversa alternativa abbiamo fatto fino in fondo quello che ritenevamo il nostro dovere. ringrazio ancora i colleghi del mio Gruppo e i colleghi dei Gruppi di opposizione. Abbiamo provato a portare avanti manovre e misure importanti; non ci siamo riusciti ed abbiamo paura che nel corso dei prossimi mesi questo Governo dovrà ritornare

*(PD)*. Signora Presidente, credo che gli italiani conoscano la gravità delle nostre condizioni e credo che sappiano che questa manovra è necessaria. Credo che le riserve e le proteste che abbiamo sentito così ampie non siano segno di irresponsabilità, né siano volte a negare i sacrifici. Penso che gli italiani vorrebbero un Governo capace di spiegare con chiarezza il senso politico e l'equità sociale delle sue decisioni. Presidente, mi scuso con lei ed anche con il sottosegretario Giorgetti, ma debbo rilevare che in altri tempi, in circostanze analoghe a queste, davanti a provvedimenti di questo peso, in Aula avremmo visto il Ministro dell'economia e l'Aula sarebbe stata presieduta dal Presidente del Senato, e con questo anche i senatori sarebbero stati presenti in maggiore numero: l'Aula oggi non trasmette al Paese il senso dell'importanza delle circostanze. Questa è una manovra biennale che vale 24 miliardi ma vista l'assoluta indeterminatezza dei risultati della lotta all'evasione e viste le incertezze sul costo delle compensazioni concordate con la Confindustria, è probabile che alla fine il risultato sia inferiore. Penso che potrebbero venire a mancare non meno di 5 o 6 miliardi di euro. Anche altri Paesi hanno promosso misure molto consistenti: la Francia, 94 miliardi in tre anni; la Gran Bretagna 48 miliardi fino al 2015; la Spagna 50 miliardi in tre anni; e la Germania, 80 miliardi fino al 2014 al 2014 (ma investirà 12 miliardi in istruzione e ricerca). I senatori del Partito Democratico hanno già ampiamente motivato le riserve sull'iniquità e la debolezza delle misure di riduzione della spesa pubblica e, per quel che riguarda le entrate, hanno indicato precise fonti alternative di gettito. Ieri, nella sua bella relazione, il senatore Giaretta ha illustrato in dettaglio una vera e propria contromanovra su fisco, spesa e sviluppo

Risulta dal dibattito, Presidente, che il Partito Democratico non teme il rigore. Abbiamo persino suggerito di elevare il valore della manovra a 30 miliardi Abbiamo suggerito di tassare le rendite finanziarie e di imporre una minima imposta ai patrimoni "scudati", che sono entrati in Italia praticamente gratis.

E anche questa volta l'assenza di misure strutturali, volte a correggere le cause dei nostri problemi, rende la manovra intrinsecamente debole. alcuna misura che possa riportare i saldi della finanza pubblica ai livelli previsti dal Patto di stabilità, mancano misure che stimolino crescita e domanda. Dal 2001, gli italiani poveri sono diventati più poveri e i più ricchi sono diventati più ricchi, e questa manovra aggrava gli squilibri, non li modera. La manovra attacca a fondo lo Stato sociale; i tagli alle Regioni colpiranno duramente trasporti pubblici locali, spese sociali, politiche ambientali, incentivi alle piccole imprese. Il Governo dovrebbe riflettere ora sulle prevedibili conseguenze per il prossimo autunno, quando si aggraverà il dramma di lavoratori e studenti pendolari, già fortemente penalizzati da una politica delle ferrovie che da una ventina di anni ha concentrato gli investimenti sull'alta velocità, totalmente trascurando le linee regionali e locali. Una manovra così concepita serve solo a prendere tempo, è un *chip* che preannuncia le misure più pesanti che il Governo sarà costretto ad emanare tra pochi mesi, già nel prossimo ottobre, con la finanziaria del 2011. 2011. Come è possibile che una maggioranza che ha un margine di 100 deputati e 50 senatori non sappia affrontare i problemi del Paese, lavori sempre in emergenza e non riesca ad approvare le leggi se non con la fiducia? Come è possibile che Berlusconi e Tremonti non vedano come il Governo stia sprofondando nello stesso abisso politico degli ultimi anni della legislatura 2001-2006? Come è possibile che non si rendano conto che il mondo è dentro quella che Alan Greenspan ha definito la peggiore crisi della storia e che l'Italia non sta affatto meglio degli altri Paesi, come sostiene allegramente Berlusconi? I motivi della cecità del presidente Berlusconi di fronte alla gravità della situazione italiana sono numerosi: tra tutti, la mancanza di senso dello Stato, l'incubo dei sondaggi e la smania di piacere e avere successo. Berlusconi non comprende che gli uomini di Stato debbono saper sfidare l'impopolarità, se i bisogni del loro Paese lo rendono necessario; ma per sfidare l'impopolarità serve coraggio politico, che è merce rara sia a Palazzo Chigi che a Palazzo Grazioli. Da poco, il presidente Berlusconi si è vantato pubblicamente - ed io non sono riuscito a sorridere, Presidente - dei successi della sua politica del cucù. La politica del cucù non gli servirà a nulla per risolvere i gravissimi problemi strutturali dell'Italia. Aggiungo solo due considerazioni di carattere politico a quanto i senatori del PD hanno già ampiamente illustrato circa le nostre posizioni. La prima questione riguarda l'atteggiamento di assoluta indifferenza del Governo nei confronti del debito pubblico, che ieri la Banca d'Italia ha comunicato avere raggiunto la cifra record di 1.827 miliardi. Come ha detto il presidente Napolitano, possiamo discutere come fare, ma non possiamo continuare a far pesare sulle spalle dei giovani un debito pubblico così spropositato. Gli interessi sul debito sono arrivati a 71 miliardi l'anno. Sono 71 miliardi bruciati, che gli italiani pagano con le loro tasse. Pensate di quanto si potrebbe ridurre la pressione fiscale se avessimo se avessimo la disponibilità di 71 miliardi l'anno! Inoltre, nessuno può garantire che nel futuro i mercati, colpiti anche dalla debolezza della nostra politica, possano imporre rialzi ai tassi. Negli ultimi anni, con i Governi del centrodestra, il valore assoluto del debito è sempre cresciuto; c'è un'evidente incapacità del Governo a contenere con misure strutturali il debito e ad incidere significativamente sui conti pubblici. Quando il ciclo di Berlusconi sarà concluso, il bilancio in termini di modernizzazione e di sviluppo del Paese sarà disastroso. Perché il Presidente del Consiglio non illustra al Parlamento quali sono le sue strategie per il rientro dal debito pubblico? Perché non dice come, con il federalismo, verrà distribuito il debito? In alcune Regioni lo Stato, indebitandosi, ha investito di più e in altre di meno, e della distribuzione del carico del debito bisognerà pur tenere conto. Perché il Presidente non spiega che cosa ha in mente? Pensa a correzioni virtuose su base annua che comportino diminuzione della spesa ed aumento delle entrate? Oppure punta solo allo sviluppo ed ha in mente un piano ambizioso di privatizzazioni e liberalizzazioni? Non chiedo al Governo di risolvere il problema del debito con questa manovra, ma di indicare la sua politica di riduzione del debito e di impegnarsi a realizzarla: questo noi dobbiamo chiederglielo formalmente. Si tratta della quarta manovra correttiva nell'ultimo anno e mezzo e non si è mai parlato di debito. Il Parlamento deve sapere, ha il diritto di sapere dove stiamo andando, e il Governo ha il dovere di far conoscere con trasparenza le politiche di breve, medio e lungo periodo sul debito. inoltre al presidente Berlusconi che il debito pubblico non si riduce con privatizzazioni tipo quelle dell'Alitalia, che invece di portare risorse nelle casse dello Stato ci è costata tra i 4 e i 5 miliardi.

e senza coscienza civile nessuna manovra, nemmeno questa, può produrre risanamento economico in un Paese malato. Il presidente Berlusconi denuncia il clima giacobino e giustizialista, ma credo che farebbe meglio a denunciare la costellazione di comitati d'affari che sta saccheggiando lo Stato italiano. Qualche anno fa, in un libro fortunato, il ministro Tremonti ha puntato il dito sulla debolezza delle regole e dei controlli. Mercati senza regole, controllori compiacenti, assenza di morale e di responsabilità: questo è il brodo di coltura delle crisi. Su tale aspetto non mi rivolgo al presidente Berlusconi, perché se so che è inutile; mi rivolgo viceversa al Ministro dell'economia: perché, ministro Tremonti, che vede tutto e comprende tutto, non ha imposto il controllo preventivo del Tesoro sulle ordinanze della Protezione civile? Perché non ha inserito nella manovra una norma per abrogare la disastrosa equiparazione dei grandi eventi alle calamità naturali, ai terremoti e alle alluvioni? Perché il ministro Tremonti non ha messo mano alle Autorità indipendenti, imponendo la nomina immediata del presidente della CONSOB e garantendo al Paese che al termine del mandato il nuovo presidente non avrà nessuna carica governativa? Se i Presidenti delle Autorità indipendenti sanno di poter aspirare a premi governativi a fine mandato, è chiaro che cessano immediatamente di essere indipendenti. Perché il ministro Tremonti consente - l'ha ricordato poco fa la senatrice Mongiello - che l'Italia venga esposta a pesanti sanzioni dell'Unione europea per proteggere chi ha violato la legge in materia di quote latte? Tutto ciò è possibile, signora Presidente, in un Paese ridotto come il nostro: due Ministri dimissionari per vicende di rilievo penale, Sottosegretari, coordinatori di partito e parlamentari del PdL indagati o colpiti da mandato di cattura. Presidente, è molto difficile dare credito a una manovra di risanamento dell'economia proposta da un Governo nel quale il proprietario della maggiore industria televisiva privata si è autonominato Ministro per la televisione.

colleghi, ho ascoltato con grande attenzione gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto in questo dibattito, a partire dal relatore. Li ho trovati interessanti, non solo per gli spunti di riflessione che se ne possono trarre, ma per il modo in cui complessivamente viene rappresentata la realtà di questa manovra. Non penso che giovi a fornire un giudizio sereno sull'azione del Governo e della maggioranza che lo sostiene l'insieme delle tante considerazioni svolte, come da ultimo quelle del senatore Zanda, che non fanno altro che gettare confusione oltre che rendere ancora più opaco il dibattito sulla manovra, che pure ha visto impegnata nei lavori della Commissione la gran parte di noi.

Eravamo partiti dal fatto che, al netto delle polemiche del gioco politico (quelle pesantemente utilizzate oggi dal senatore Zanda), anche l'opposizione guardava in termini non ostativi

Mi ha colpito di più il rammarico del presidente Marini, al quale vorrei provare a rispondere. Per questo parto necessariamente dai fatti che determinano il contesto in cui il Governo è costretto a muoversi e che lo obbligano a varare il provvedimento che stiamo discutendo. La congiuntura negativa ha delineato un contesto - e su questo penso siamo tutti concordi - certamente più complesso di quello che possiamo descrivere nel poco tempo che ci viene concesso Le tensioni che la crisi ha provocato nella finanza prima e nell'economia reale poi si stanno spostando sui conti pubblici: il rischio di *default* non è confinato alla sola Grecia, come tutti sanno, ma può propagarsi; le tensioni speculative in agguato in molti Paesi (leggiamo in queste ultime ore le notizie relative ai rischi del Portogallo) continuano a preoccupare commentatori, economisti ed autorità politiche e dovrebbero preoccupare anche noi. Fronteggiare tali rischi, contenerli e reinnestare un circolo virtuoso di crescita è ancora possibile, a patto che si intervenga significativamente sui conti pubblici: sul *deficit*, che deve dimagrire

innanzi tutto con un contenimento strutturale della spesa pubblica. La pensa così anche l'Europa, che il 12 maggio scorso ha deciso un'operazione comune o meglio - vorrei sperare - condivisa dai Paesi membri, per adottare manovre di rientro da ingenti disavanzi pubblici. Ora, se questo è il contesto, qual è il giudizio sull'azione intrapresa dal Governo? In sintesi, credo che l'azione dell'Esecutivo sia stata improntata ad un sano realismo, un sano realismo, lontano da atteggiamenti di retroguardia (come qualcuno aveva paventato), ma anche da inutili fughe in avanti. È in questo modo che ritengo vada letta la manovra oggi al nostro esame. Tale manovra sta all'interno di obblighi assunti in sede europea.

dal governatore Draghi nella sua relazione annuale, dall'Europa: è di ieri la notizia del significativo apprezzamento che l'Unione europea (in particolare, l'ECOFIN) ha espresso sui contenuti,

E aggiungerei, aspetto non secondario, diversa da quelle che stanno compiendo altri Paesi, sia per la quantità che per la qualità delle azioni intraprese, che io considero migliori, nell'ottica di contenere le misure più aspre (quando parliamo di tagli, parliamo di misure aspre) ed evitare ricadute oltremodo negative sui redditi e sui consumi. per rispondere alla capogruppo Finocchiaro, che proprio ieri paventava i rischi depressivi di questa manovra sul risparmio e sui consumi. Da un lato c'è il contenimento delle spese, la riduzione significativa del rapporto tra spesa pubblica -essenzialmente quella corrente, certo - e il PIL. Desidero ricordare un dato di ordine quantitativo, tanto per avere un ordine di grandezza delle cose di cui parliamo: nel 2009 la spesa finale delle pubbliche amministrazioni è stata di circa 800 miliardi di euro, oltre il 52 per

Da questo punto di vista, mi sembra che il Governo abbia ben presente che la via del risanamento dei conti pubblici passa da alcuni settori centrali per l'intera economia pubblica: impiego, sanità e pensioni. Intervenire su tali settori certamente non esaurisce gli spazi di manovra: penso, ad esempio, al tema a me caro dei consumi intermedi, sviluppato molte volte in quest'Aula dal senatore Baldassarri, sui quali appare possibile un deciso intervento di razionalizzazione, non solo sull'entità complessiva, ma soprattutto sulle modalità operative che ancora determinano la formazione e la crescita indesiderata di questa spesa. Certo, rimane ancora aperta la questione del concorso al risanamento da parte delle Regioni, ma siamo convinti che il punto di equilibrio possa essere trovato in sede di applicazione di quel federalismo fiscale al quale in tanti stiamo lavorando. L'altro pilastro su cui si basa la manovra è, inevitabilmente, l'acquisizione di nuove risorse: in altre parole, la lotta all'evasione fiscale. Non è realistico, infatti, pensare che il blocco dei contratti pubblici o la lotta ai falsi invalidi consentano di recuperare 25 miliardi di euro: lo sapevamo già. È necessario il contrasto a fenomeni di evasione, che apporterà circa 20 miliardi di euro nei triennio 2010-2012. A parte le polemiche sulle attività di contrasto «alla Visco», sulle quali, vorrei ricordarlo ancora una volta, siamo idealmente lontani - molto lontani - ricordo che la lotta all'evasione va condotta proprio con il redditometro e con il conto IVA conosciuto dal fisco in tempo reale. Non credo che, come dice il senatore Rossi, che leggo sempre con molto interesse, il Ministro dell'economia finirà col fare quello che fanno tutti i Governi, cioè aumentare la pressione fiscale. Anche qui, la nostra visione della società e dell'economia è diversa, molto diversa. Ricordo che il Governo Prodi aumentò di due punti la pressione fiscale, ben prima della grave crisi finanziaria che il nostro pianeta sta vivendo. il taglio della spesa pubblica e il recupero di risorse da redditi oggi non conosciuti, in prospettiva significano per noi la riduzione delle aliquote fiscali. L'innalzamento dell'età pensionabile delle donne nella pubblica amministrazione per noi non è solo un modo per fare cassa, ma costituisce, e mi auguro costituisca sempre di più, anche

come ha ricordato il sottosegretario Casero durante la discussione in Commissione, da quello per così dire particolare non mancano significativi spunti di riflessione. L'*iter* in Commissione - e spero sia apprezzato il fatto che il testo sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia sia assolutamente aderente al dibattito al dibattito svolto in quella sede - non solo non ha «spolpato» il provvedimento, ma ha consentito di migliorare, anche grazie al contributo dei colleghi dell'opposizione, quei punti per i quali lo stesso Esecutivo si era dichiarato disponibile al dialogo. A parte il riconoscimento di indubbie istanze di equità (penso alla questione delle invalidità, al settore sicurezza, a quello della scuola, dove affluiscono risorse per la valorizzazione e la professionalità dei docenti), non sembrano di poco conto, ad esempio, le modifiche introdotte al pacchetto fiscale, dalla compensazione dei crediti della pubblica amministrazione, all'esecutività posticipata dell'accertamento, al regime fiscale di attrazione europea. Peraltro, come non ricordare le ripercussioni favorevoli sull'economia e la vita di alcuni territori derivanti dalla possibilità di sbloccare i fondi per la realizzazione di importanti opere infrastrutturali? Penso solo alle rafforzate garanzie di finanziamento per la realizzazione della galleria del Brennero. E questo, poi, non ha impatti positivi sullo sviluppo? E non ha rilevanza strutturale? Potrei continuare nell'elenco. Arriverei a confutare l'adagio, evocato qualche giorno fa da un autorevole ed esperto commentatore, Mario per cui il maligno si nasconde nei dettagli. Al contrario, questa manovra, salvaguardata nei saldi e nell'impianto generale, forte di norme strutturali sul contenimento della spesa pubblica e dei miglioramenti apportati in Commissione e in quest'Aula che l'hanno rafforzata, ci è riconosciuta dall'Europa come una delle migliori tra le iniziative intraprese dai Governi dei Paesi membri e al presidente Berlusconi va il merito di averla voluta e sostenuta. *(Applausi della senatrice Colli).* PRESIDENTE. È iscritta

tre novità e tre criticità: tre novità che purtroppo, nel corso del dibattito, sono state dimezzate, e tre criticità che purtroppo, nel corso del dibattito, si sono rafforzate. Le tre novità dimezzate consistono sostanzialmente nel fatto che per la prima volta si riconosce che c'è una crisi, per la prima volta si parla sostanzialmente di tagli di spesa, per la prima volta si fanno i conti reali con l'evasione fiscale.

Noi siamo entrati nella recessione decisamente con il fiato corto. Lo abbiamo già detto ed io personalmente l'ho fatto presente più volte in quest'Aula. Un Paese che ha visto la caduta del reddito *pro capite* dal 2000 al 2009 del 4,1 per cento è un Paese che sta diventando più povero lo sta diventando perché l'andamento della produttività in Italia è da troppo tempo assolutamente insoddisfacente. Questo significa che la nostra economia non è più in grado di generare reddito futuro, e questa è una sciagura perché si può essere temporaneamente deboli, si può essere temporaneamente più poveri, ma noi lo stiamo diventando strutturalmente. Non è più un problema contingente, il nostro: il nostro, ormai, è oggettivamente un problema strutturale, nei confronti del quale non si stanno mettendo in essere delle contromisure strutturali e non lo si sta facendo da troppo tempo. C'è una ostinata persistenza della nostra criticità e una ostinata persistenza a non affrontare i punti nodali della nostra debolezza congiunturale. Esistono macroscopici squilibri nel nostro Paese su cui non stiamo intervenendo, se non nei dibattiti e nella comune condivisione della della loro identificazione, e c'è una incapacità ad individuare, invece, gli interventi che possono portare al loro superamento. Parlo di macroscopici squilibri che sono di genere.

è diventato enorme e questo è ancora più grave se consideriamo le grandi risorse economiche che sono state impiegate per ottenere un risultato di questa natura. Quindi, c'è un problema strutturale che riconosciamo in tutti i dibattiti, nei confronti del quale stiamo facendo, anche con questa manovra, assolutamente poco. Il taglio delle spese. Credo che il taglio delle spese sia, così l'avevo letto all'inizio nella manovra, sostanzialmente una delle vere novità di cambio di tendenza. Letti gli atti, però, devo riconoscere che quanto detto stamattina dal collega senatore professor Baldassarri in ordine alla percezione reale del dato di spesa e al calcolo effettivo

che ricorda per certi aspetti un po' quel che capita, in misura molto minore, con gli autovelox nei comuni. Si usano cioè degli strumenti per fare cassa, anziché per ispirare una cultura diversa. Qui mi pare che stiamo facendo la stessa cosa. Perché? Perché la lotta all'evasione fiscale in un Paese in cui l'evasione è endemica deve avere una prospettiva di lungo periodo. Le cattive abitudini non si buttano dalle scale, ma si fanno scendere

e che credo siano invece da tenere in debito conto, perché questa manovra è fatta non solo per l'opinione del Paese, ma anche per l'opinione dell'Europa, dell'Europa, delle agenzie di *rating* e degli investitori istituzionali. Altrimenti, tanta durezza, non sarebbe neanche comprensibile. Da questa manovra esce un'immagine del Paese che peserà sul nostro futuro. Quindi, i conti dovranno quadrare e la previsione di un PIL al 2 per cento nel 2012 per farci rientrare nel Patto di stabilità, stante la delicatezza dei dati su cui si fonda, è del tutto difficile da mantenere.

sul fatto che stiamo utilizzando un risparmio accumulato dalla mia generazione e da quella che mi ha preceduto, mentre abbiamo di fronte a noi generazioni che non sono in condizione di ripristinare tale risparmio, non sono in condizione di mettere insieme quello che oggi stiamo mangiando per reggere alla crisi. Al riguardo bisogna intervenire.

Noi, in verità, abbiamo fatto, per ore ed ore, in Commissione, un esercizio autistico, perché non siamo riusciti a trovare un punto comune nell'interesse generale. Signora Presidente, questa manovra economica, che fin dall'inizio abbiamo giudicato negativamente per il suo tratto di iniquità innanzitutto, è stata in realtà peggiorata nel corso dell'esame in Senato, né viene migliorata dal maxiemendamento del Governo che corregge soltanto alcuni aspetti marginali. Una manovra di correzione dei conti pubblici italiani, lo abbiamo detto, era certamente necessaria per ragioni interne e di rapporto con l'Europa e poteva rappresentare l'occasione per chiamare tutto il Paese ad un cimento straordinario; come si sa, gli italiani sono capaci di gettare il cuore oltre l'ostacolo di fronte alle grandi difficoltà e alle sfide più impegnative. Per fare questo servivano però alcune cose: una visione unificante del Paese e la scelta di dialogare con le opposizioni, un principio di equità nella ripartizione dei sacrifici, un'idea della crescita capace di liberare le energie vitali e imprenditoriali del Paese e, soprattutto, di indicare una prospettiva, una speranza alle giovani generazioni, al Sud, alle donne, a chi ha perso il lavoro. Tutto questo non c'è stato e non c'è. Al contrario, le parole del *Premier* e quelle del ministro Tremonti sono state tutte nel segno della divisione del Paese e del mantenimento dello *status* *quo*. Il Ministro dell'economia inoltre ha esternato ad alta voce il suo personale convincimento, che palesemente ispira la manovra stessa: considerato che sotto il Garigliano gli italiani sono prevalentemente dei cialtroni, è bene che il Sud paghi il prezzo più alto. Il simbolo di questa determinazione è rappresentato dall'emendamento fatto approvare in Commissione a favore dei 67 allevatori del Nord, tanto cari alla Lega, che ancora oggi non hanno pagato la multa sulle quote latte. Un emendamento palesemente scoperto sotto il profilo delle risorse, anche perché non considera l'infrazione e la sanzione già annunciata dalla Commissione europea e si pregia, tra l'altro, di occultare le pesanti sanzioni già pagate lo scorso anno con i fondi FAS per condonare l'evasione delle multe sulle quote latte di altri allevatori del Nord, per un importo vicino al miliardo di euro sottratto al Mezzogiorno. Un premio ai più disonesti - quello di oggi - ed un altro schiaffo al Sud nel silenzio veramente sconcertante di tutti, dico tutti, i senatori meridionali del Partito della Libertà. Sarà stata forse l'enormità di questa scelta ad aver ispirato il successivo emendamento - si sa, dopo il bastone viene la carota - verso gli elettori del PdL con il rifinanziamento dei 25.000 lavoratori socialmente utile della sola Sicilia, in barba al rigore della manovra sulla spesa e a tanti altri migliaia di LSU meridionali. Con gli interventi dei senatori del Partito Democratico in Commissione bilancio abbiamo dimostrato che sarebbe stata possibile un'altra manovra, diversa da quella presentata dal Governo. Questa è una manovra che esaspera gli squilibri territoriali e sociali, che colpisce i lavoratori pubblici ed i redditi più bassi e che impone alle Regioni pesanti limitazioni sui servizi essenziali per i cittadini attraverso un taglio dei trasferimenti senza precedenti. Sono stati non più di una ventina gli emendamenti veramente significativi della contromanovra del Partito Democratico lungo le direttrici dell'equità, della crescita e delle riforme strutturali. Noi consideriamo che una profonda ristrutturazione della macchina pubblica è certamente la via maestra per una più forte riduzione della spesa corrente, tale da consentire tagli reali sugli sprechi e le improduttività. una via di riforma e non intervenire, come si sta facendo con le manovre degli ultimi due anni, attraverso i cosiddetti tagli lineari, che ottengono solo lo scopo di peggiorare la qualità del lavoro e dell'offerta di servizi ai cittadini. Nonostante il chiaro profilo dei nostri emendamenti, non vi è stata nessuna interlocuzione del Governo con le proposte del Partito Democratico e delle opposizioni. D'altra parte, la Commissione bilancio ha vagliato e votato oltre 1.200 emendamenti della sola maggioranza, a riprova delle tensioni interne e della pressione di vari gruppi di interesse che hanno condizionato in maniera significativa il testo finale. Quote latte, LSU solo per la Sicilia, ripristino per molte società ed enti pubblici di compensi vari a sindaci, revisori, consigli di amministrazione, dimostrano una disponibilità sul fronte della spesa senza sapere poi incidere effettivamente sulla qualità e sulla struttura. Ad essere incerta è anche l'entità delle nuove entrate, quelle della lotta all'evasione, che appare sovrastimata, ma soprattutto sconfessata dalla stessa vicenda delle quote latte, che lascia aperta la via a nuovi, futuri, probabili condoni di vario genere. Sono molti a ritenere che presto verrà in luce la necessità di una nuova manovra che darà luogo a pesanti ed ulteriori tagli. Ma come senatrice del Meridione d'Italia voglio dire che con questa manovra il Governo volta platealmente le spalle al Sud a vantaggio del Nord. Con gli emendamenti che ho sostenuto e con questo intervento voglio invece dare la parola al Sud dei giovani, delle donne, degli amministratori onesti (che sono la maggioranza e sono di centrodestra e di centrosinistra e andrebbero sostenuti e non umiliati invece come si continua a fare in anche perché quando finiscono gli amministratori onesti fuori resta la criminalità e la camorra), al mondo della scuola, della ricerca e della cultura, ai cassaintegrati, ai precari e ai più svantaggiati, tra cui in alle lavoratrici pubbliche, che dovranno andare in pensione a 65 anni in omaggio ad un'idea di parità quanto meno poco fantasiosa. Che fine hanno fatto gli impegni elettorali per un piano straordinario per il Sud e quelli per il credito, con la tanto propagandata Banca per il Mezzogiorno? Tutti gli emendamenti da noi presentati sono stati respinti: quello sugli istituti di ricerca e cultura, sull'adozione di ricercatori per le università meridionali, sulle detrazioni fiscali per le donne e per la cura dei bambini e degli anziani, sulla possibilità di scegliere l'età della pensione tra 62 e 68 anni

che cancellano tutte le delibere di spesa degli ultimi dieci mesi dopo la decisione, pubblica e discussa, di fuoriuscire dal Patto di stabilità, a fronte di una crisi drammatica e su richiesta di tante ed associazioni di impresa; una possibilità - quella di fuoriuscire dal Patto di stabilità - che questa manovra riconosce - chissà perché - solo a Roma. E ancora è stato respinto l'emendamento che consentiva di far vivere le zone franche urbane, che con questa manovra saranno definitivamente cancellate e sostituite con aree cosiddette a burocrazia zero, che affidano a sindaci e prefetti la responsabilità di elargire, direttamente e discrezionalmente, gli incentivi alle imprese, con l'unica eccezione, a questo punto veramente importante - lo diceva il senatore Marini - della città dell'Aquila. Io mi batto con foga su questo tema. Infatti, non si capisce perché dopo l'individuazione delle 22 zone franche urbane, 18 delle quali nel Mezzogiorno, e finalmente dopo l'approvazione della Commissione europea, non si è andati avanti, mentre si poteva finalmente sperimentare quel sistema innovativo di fiscalità di vantaggio automatico per le zone svantaggiate, fortemente voluto da tante imprese meridionali, sul modello di esperienze già realizzate in Francia con successo, che avrebbe potuto chiudere definitivamente la stagione degli incentivi e avviare una nuova positiva esperienza di sviluppo dal basso tutta centrata sull'imprenditorialità il capitale sociale, piuttosto che sul sussidio statale. Investire sulle zone franche urbane sarebbe stato un segnale positivo a quel Sud che non si lamenta, ma che è ancora una volta pronto a rimboccarsi le maniche. A questo punto non mi resta che citare l'unico obiettivo raggiunto, quello che riporta al 74 per cento la percentuale di accertamento di invalidità per ottenere l'indennizzo, in cambio giustamente di più rigorosi controlli, e quello che prevede il ritiro dell'emendamento più incivile, che avrebbe eliminato la soglia di 20 per la formazione delle classi con alunni con disabilità. Più che di una vittoria, si tratta soltanto di un barlume di buon senso della maggioranza, in un contesto che purtroppo resta profondamente negativo in una manovra che moltiplica le ingiustizie.

e la sua sostituzione - non è una definizione mia - con provvedimenti *light* pressoché immodificabili. L'annuncio doveva mettere la parola fine a quell'andazzo che vedeva il Governo produrre un testo sul quale poi si scatenava quello che il Ministro definì l'assalto alla diligenza. Invece, con la consueta disinvoltura il Governo e la sua maggioranza, facendo finta di nulla, hanno ripercorso gli stessi riti che spudoratamente un anno fa avevano dichiarato conclusi. D'altra parte, non è una novità. Il Capo del Governo, con leggiadra spudoratezza, passa da annunci roboanti sulla fine della crisi, sul fatto che la crisi è solo psicologica e che tutto si risolverebbe spargendo ottimismo e convincendo gli italiani a spendere di più, spendere di più, a supponenti dichiarazioni sulla sostenibilità dei conti, sul fatto che non si mettono le mani nelle tasche degli italiani, per poi produrre provvedimenti che direttamente o indirettamente fanno raggiungere nuovi record assoluti alla pressione fiscale. Ma per ora il *Premier* può stare tranquillo: gli esiti della manovra faranno spendere di più gli italiani. Spenderanno di più i pendolari ai caselli autostradali, le famiglie, che spenderanno di più per le tasse e le tariffe locali per asili nido, mense scolastiche, trasporti e sanità. Siamo poi in attesa di conoscere l'applicazione dell'annunciata tassa comunale sugli immobili e temo che anche in questo caso avremo amare sorprese. La verità è che il vostro Governo ha ricevuto in eredità un debito pubblico al 103,5 per cento del PIL e lo ha portato al 118 per cento, più o meno come la Grecia. La pressione fiscale è al 43,2 per cento - mi spiace che la senatrice Bonfrisco sia appena uscita: forse non voleva sentirsi ricordare questi dati - un vero primato, che fa onore all'uomo dello slogan «meno tasse per tutti», e, per la prima volta da quasi vent'anni, è stato azzerato l'avanzo primario. Altri colleghi prima di me, in particolare il relatore di minoranza Giaretta, hanno evidenziato come il Paese si sia indebolito nel corso di questi anni. I dati sul PIL e sulla competitività, la perdita di produttività parlano chiaro. Su un dato però voglio soffermarmi un momento, quello della disoccupazione giovanile che oggi nel nostro Paese è circa al 30 per cento. Siamo di fronte ad un dato drammatico, con un Governo che non ritiene di doversi impegnare in alcuna politica adeguata per combattere questa che è una vera piaga. Un Paese governato in questo modo è un Paese che non sa investire sul suo futuro, destinato a veder sprofondare i giovani e le famiglie in quell'atteggiamento depresso, tante volte deprecato dal *Premier,* che colpisce tutti coloro che non intravedono un futuro. E non è vero che non si poteva fare altro, si potevano fare scelte differenti: le abbiamo sollecitate, ma siamo rimasti inascoltati. Voglio ricordarne qualcuna. Si poteva inasprire il prelievo fiscale sui capitali regolarizzati attraverso lo scudo fiscale: sarebbe stata una misura di equità. Il nostro Paese ha consentito un'operazione con un'aliquota scandalosamente bassa: nessun Paese europeo che ha fatto questa scelta ha applicato aliquote del genere. Sarebbe stato necessario cominciare a rivedere il rapporto tra la tassazione sulle rendite finanziarie e quella sul lavoro dipendente, che nel nostro Paese ed è più basso di tutti i Paesi europei. Se è vero che sono necessari tagli alla spesa pubblica, è altresì vero che poco credibile è una riduzione che all'80 per cento colpisce le amministrazioni locali e solo per il 20 per Si sarebbe potuto intervenire in maniera più equilibrata; scaricare i tagli sugli Enti erogatori di servizi provocherà sicuramente un aumento delle tariffe a carico dei cittadini. Ci sarebbe poi voluto più coraggio sulla politica della casa, l'abbiamo invocato diverse volte: la tassazione secca al 20 per cento accompagnata dalla detrazione del 20 per cento per la spesa per l'affitto da parte degli inquilini. È evidente; la spesa iniziale non è da poco, non sarebbe stata indifferente, ma sicuramente sarebbe stata compensata con una notevole emersione di nero ed un diffuso stimolo per l'economia. Il Governo sta invece varando una finanziaria - credo sia opportuno continuare a chiamarla così - senza slancio, senza sguardo al futuro, senza prospettive di crescita. Un provvedimento che non raggiungerà l'obiettivo di sistemare i conti e che invece raggiungerà il risultato di far pagare di più i cittadini e deprimere ulteriormente le prospettive di crescita. Lo fa inoltre nel modo peggiore. Un anno fa si era deciso di riformare la legge finanziaria per evitare l'assalto alla diligenza. Dopo i proclami concludiamo queste giornate passando dall'assalto alla diligenza al mercato delle vacche. Il Governo infatti, ostaggio della Lega, sospende il pagamento delle quote latte. Ad ognuno il suo. Ogni pezzo della maggioranza incassa prebende. Chi continua a favorire gli evasori, chi i disonesti delle quote latte, ognuno cioè trova qualche cosa per il nocciolo duro del suo elettorato. Intanto i cittadini, soprattutto quelli che vivono del proprio lavoro, pagano per tutti. Così non si può andare avanti. Noi diciamo no alla fiducia al Governo, che è un no alla legge finanziaria spacciata per decreto. Un no ad una politica economica che non garantisce un futuro al nostro Paese, un no ad una maggioranza che invece di dedicarsi ai problemi degli italiani impegna la maggior parte del suo tempo a discutere delle proprie divisioni, dei problemi del suo capo e di quelli dei suoi accoliti. Un no, signor Presidente, per rilanciare una speranza ed una politica diversa per tutti.

Morando e Giaretta, fra gli altri, mi induce a concentrare il mio intervento sulla questione della ricostruzione del *post* sisma abruzzese. Dopo più di 15 mesi dal terremoto gli aquilani scoprono di essere stati abbandonati: nessuno ha più sotto controllo la situazione. Ordinanze illeggibili hanno creato una grande confusione; ci sono imprese quasi sul lastrico perché non vengono pagati i lavori effettuati nell'emergenza, commercianti che non sanno se e quando potranno riaprire i loro negozi, migliaia di persone in cassa integrazione che non ricevono nemmeno quel reddito sociale che per molti è diventata l'autonoma sistemazione. Un quadro che definire sconfortante è poco. Quello che inquieta è che anche la classe politica al Governo del Paese e della Regione è allo sbando. Parlamentari e amministratori che sbattono la porta dicendo di non voler essere complici di un Governo che vuole punire, non si sa bene perché, L'Aquila e gli abitanti del cratere. Un Sindaco che addirittura si appella ai direttori dei giornali nazionali perché nei palazzi romani non sa più a quale Ministro votarsi. E poi il Presidente della Regione, il commissario di Governo, che va a Roma tre volte alla settimana per sentirsi rispondere, nelle segreterie dei Ministeri, che non c'è un euro da spendere. Gli unici che hanno un po' le idee chiare sono forse i Sindaci dei piccoli Comuni del cratere che per dimensione sono più facilmente gestibili: fra mille complicazioni hanno messo a punto perimetrazioni, piani di recupero, organizzato aggregati e consorzi. Uno di loro pochi giorni ha fatto una stima dei danni secondo la quale se domattina arrivassero i soldi necessari ricostruirebbero tutto in tre anni. Però i Sindaci (piccoli o grandi) nessuno li sente e sono costretti a fare la fila per pietire un incontro con burocrati che spesso ne sanno meno di loro. Un quotidiano nazionale ha reso noto lo scempio di un palazzo storico dell'Aquila, signora Presidente, dove ci sono affreschi bucati per far passare i cavi di messa in sicurezza dell'edificio. Ma basta farsi un giro sia dentro la città che nell'immediato circondario per vedere chiese storiche, fra le più belle d'Abruzzo, che stanno cadendo a pezzi. Si sono spesi milioni di euro per puntellare case che andranno abbattute, mentre i monumenti, quelli veri, sono lì ad aspettare che la loro sorte venga segnata definitivamente. All'Aquila servono (come è accaduto per Friuli, Irpinia e Umbria) norme chiare e flusso certo di fondi; altrimenti, quei pochi soldi che arriveranno finiranno nelle tasche di soliti noti e, quel che è peggio, L'Aquila non sarà ricostruita. Gli aquilani sono scesi in piazza, compatti, per urlare a tutta Italia il proprio dramma: «Salvateci, perché stiamo morendo». Mentre l'Italia tutta è convinta che il miracolo berlusconiano sia perfettamente riuscito, all'Aquila si combatte ogni giorno per far partire una ricostruzione ancora in alto mare, per tamponare una disoccupazione dilagante. Insomma, il *gap* fra la realtà abruzzese e la *fiction* mediatico-governativa è clamoroso, pari, forse, solo al diverso trattamento che la stampa ha riservato a Napoli e Palermo per l'emergenza immondizia. Al di là delle polemiche sulla copertura mediatica, la vicenda aquilana dimostra ancora una volta lo spregiudicato *modus operandi* di questo Governo: un Esecutivo che è ben felice di passare le proprie funzioni o, meglio, i propri doveri agli enti locali, salvo poi dimenticarsi di trasferire anche le risorse finanziarie necessarie. L'eliminazione dell'ICI con la contestuale riduzione dei fondi trasferiti ai Comuni e i tagli dell'ultima manovra nei confronti delle Regioni sono due precedenti abbastanza emblematici, con la differenza però che l'economia aquilana è in ginocchio e difficilmente potrà reggere al «ponziopilatismo» governativo. Da quando, a gennaio 2010, la Protezione civile ha passato la «patata bollente» al governatore Chiodi e al sindaco Cialente, i fondi statali hanno cominciato a scarseggiare: ormai ne arrivano pochi e con grave ritardo. I risultati, signora Presidente e signor rappresentante del Governo, sono sotto gli occhi di tutti: la ricostruzione delle case poco danneggiate stenta a partire perché i finanziamenti pubblici languono e le imprese che hanno iniziato i lavori sono andate in crisi di liquidità perché gli avanzamenti nei lavori non vengono pagati; ci sono 4.000 aquilani ancora negli hotel, da sommare ai 30.000 che prendono il contributo di sistemazione autonoma e che sono fuori dal proprio Comune e dalla propria casa; 16.000 disoccupati non vedono futuro, visto che le poche imprese che ancora lavorano faticano a farsi pagare. una situazione drammatica nella quale il ministro Tremonti non s'era fatto scrupolo di assestare il colpo di grazia: stando al testo iniziale della manovra, dal 1° luglio prossimo, nelle zone colpite dal sisma, si sarebbe ricominciato a pagare ogni imposta, salvo che per pochi soggetti. Ma è quella di martedì 6 luglio una pagina nera che verrà ricordata con altrettanto dolore, ma forse con più rabbia, di quella che un anno fa ha distrutto migliaia di vite. Dopo il danno c'era da ricostruire, aiutare, incoraggiare, motivare e invece è arrivata la beffa. A distanza di un anno, sono arrivati a Roma, con pullman, macchine e treni, i sopravvissuti alla tragedia aquilana per manifestare e ricordare pacificamente alle istituzioni e al Governo di avere pazienza ancora, di rimandare l'avvio delle restituzione delle imposte sospese, l'avvio del pagamento di quelle ordinarie, per non soffocare di debiti per pagare le tasse. Erano venuti a chiedere giustizia, non pietà, per chi ormai da oltre un anno non ha più nulla. Sono la testimonianza vivente di quanto ancora c'è da fare per quelle terre, di quanto il Governo abbia pasciuto quei cittadini solo di promesse per poi abbandonarli dicendo al Paese che si era già fatto tutto. In 5.000 hanno lanciato con forza, per l'ennesima volta, un grido per la sospensione delle tasse, l'occupazione, il sostegno all'economia; senza bandiere o striscioni di partito, ma con solo due colori predominanti - il verde (della speranza)

Si sono ritrovati a piazza Venezia, nel centro della capitale, a manifestare contro le stesse persone che avevano promesso loro di restituire loro i diritti, contro quegli angeli che un anno prima, tra le macerie, avevano faticato, pianto e sperato con loro per recuperare ciò che era rimasto, per estrarre i corpi dei loro figli, familiari, amici. La mancanza di politica, di dialogo, di collaborazione ha fatto sì che quegli stessi uomini, con gli stessi simboli sui cappelli e le loro divise abbiano malmenato e spintonato, creando terrore e sgomento tra i cordoni dei manifestanti inermi. Senza che nessuno in quella situazione abbia pensato alle conseguenze o agli effetti sugli animi di chi stava protestando perché senza lavoro, senza casa, senza qualche figlio, o parente, o amico, perché deceduto. E a continuare a non sapere nulla della ricostruzione. Non credo ci sia rimasto altro che piangere per un Governo come quello Berlusconi, che trova i soldi per inventarsi un nuovo Ministero e nuovi privilegi di casta e dimentica di sostenere nella speranza di ripartire un popolo fiero che ha dato tanto. Sono serviti i manganelli per far cambiare idea a Palazzo Chigi: oggi, nel testo del maxiemendamento, signor Sottosegretario, leggiamo che le tasse verranno restituite in 10 anni come il Partito Democratico vi sta chiedendo da 15 mesi, di farlo insieme, non solo noi - ma senza alcuno sconto, come invece è avvenuto per i terremoti di Umbria, Marche e Molise e per il dramma di Messina, come voi sapete. Si chiede solo, eguale dignità, come chiedono gli abruzzesi che vivono fuori dal cratere, che hanno visto danneggiate case, scuole, ospedali, chiese, ma che hanno la colpa di aver subito una scossa inferiore al sesto grado, e per questa colpa non avranno alcun tipo di risarcimento. Avranno ancora gli italiani, anche nella lunga era Berlusconi, diritto di essere considerati eguali, indipendentemente dalla Regione nella quale sono residenti? Il ministro Maroni, non l'opposizione, nell'immediatezza del dramma, due giorni dopo - lo può verificare, signora Presidente - affermò che per la ricostruzione sarebbero occorsi non meno di 13-15 miliardi di euro. Qualcuno del Governo o della maggioranza ha mai dimostrato il contrario? E allora, perché su questo argomento il Governo fa finta di non capire? Perché la maggioranza si stressa quando ve lo ricordiamo? La gente può abituarsi, ma non dimentica, e dopo le tante promesse arriverà a chiedere il conto anche a voi, come lo ha chiesto a noi, e lo abbiamo pagato caro, quel conto. Sarà quello il momento nel quale vi chiederanno: dopo l'emergenza, passati anni, perché non avete ricostruito? A quel punto tutto il *bluff* verrà allo scoperto, e le grandi bugie raccontate agli italiani dalla crisi che non c'era, agli abruzzesi che già stanno tutti a casa - si rovesceranno a valanga su di voi e vi seppelliranno, ma senza ridere di questo nuovo dramma!

n. 533, nonché del parere della Giunta per il Regolamento espresso nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Campania a seguito delle dimissioni del senatore Sergio Vetrella, ha riscontrato, nella seduta odierna, che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva il predetto senatore è Franco Cardiello. Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e proclamo senatore Franco Cardiello.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, signor relatore presidente della Commissione bilancio, innanzi tutto vorrei collegarmi alla commozione comprensibile e giusta del collega Lusi,

e così ci rimette chi non dovrebbe rimetterci, non per responsabilità sua o delle forze dell'ordine che intervengono, ma per elementi assolutamente estranei a queste vicende. In uno Stato democratico, a volte sono questi i prezzi che si devono pagare per una libertà che è sovrana,

Ora stiamo intervenendo per il rafforzamento e la stabilizzazione del sistema finanziario pubblico interno e per fare ripartire la competitività economica. Ricordiamo che questa manovra contrasta anche con decisione l'evasione fiscale. La Commissione ha lavorato con impegno e responsabilità sul decreto del Governo, ben articolato e completo, apportando significative integrazioni e miglioramenti, come è stato riconosciuto dal ministro Tremonti. Di questo apprezzamento siamo ovviamente compiaciuti. Facciamo alcuni esempi di argomenti vicini alla gente che hanno trovato posto in questo provvedimento. Per la tracciabilità dei pagamenti, l'uso dei contanti è limitato a 5.000 euro e andranno comunicate all'Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di valore non inferiore a 3.000 euro.

Non è solo un cambiamento di sigle, ma una vera e propria rivoluzione amministrativa, ove ora il cittadino è al centro del sistema. Ci siamo impegnati per evitare la possibilità di alcune forzature nei settori della cittadinanza, della residenza e della sicurezza: su questi siamo intervenuti ed interverremo ancora in futuro, se sarà necessario. norme e requisiti nuovi per le pensioni, specialmente nel settore pubblico, per garantire un futuro sicuro, soprattutto per le nuove generazioni che entrano nel mondo del lavoro:

regole più stringenti per i rogiti, contro gli abusi; nelle compravendite immobiliari, le parti dovranno dichiarare la conformità delle planimetrie alla situazione reale ed il notaio dovrà conformare i dati dei registri con quelli catastali. Abbiamo lavorato in Commissione con decisione, ottenendo significativi risultati in tema di disabili, sicurezza, enti locali, infrastrutture territoriali ed agricoltori.

per tutto il nostro territorio. Per questo siamo orgogliosi di esserci sporcati i piedi e le mani anche in questo settore e siamo grati al relatore ed al Governo di aver compreso il valore delle nostre proposte e di averle accolte. Questa manovra è equamente suddivisa sulla contrazione della spesa pubblica centrale e degli enti locali. Le Regioni hanno fatto sentire voci di contrarietà, ma in realtà non tutte. Parliamo allora degli sprechi che ci sono stati nelle Regioni. Facciamo alcuni esempi, partendo dal Lazio. La nuova governatrice Polverini ha ricevuto in eredità dalla Giunta Marrazzo un *deficit* nella sanità di 1,3 miliardi di euro (un terzo dell'intero *deficit* nazionale, che è pari a 3,4 miliardi), ma, con competenza ed impegno, nelle prime settimane, ha già individuato circa 200 milioni di risparmi strutturali, senza far scendere il livello delle prestazioni erogate. Quindi, se si vuole, si può risparmiare. La Guardia di finanza ha contestato una maggiore spesa per acquisto di farmaci, dal 2004 al 2006, di circa 250 milioni. Nel 2009, quella Giunta ha dato 400.000 euro per finanziare un centro di cinematografia in Marocco:

euro, accorgendosi poi che i mezzi erano troppo larghi per entrare in deposito. Per finire, passiamo alla Sicilia: basta dire che viene fatta una TAC ogni 56.000 abitanti, quindi più che in Emilia o in Toscana. Solo che nelle Regioni del Centro-Nord i tempi di attesa sono circa 28 giorni

rischio e conti con l'esterno delle regioni italiane», a cura di Paolo Savona ed altri autori, ha rafforzato la necessità di questa manovra, vista non come punto di arrivo, ma di partenza verso il federalismo.

A questa manovra avrei voluto presentare un emendamento, alla luce della disfatta degli azzurri nei campionati mondiali di calcio in Sudafrica. Essere andati a casa, oltretutto nel modo peggiore della storia, ci costa circa 50 milioni di dollari andati in fumo: dai 5 ai 21 milioni di mancati premi FIFA una trentina di milioni di minori introiti tra *sponsor* e fornitori. Torniamo comunque a casa con 9 milioni (1 milione come partecipazione e 8 milioni per aver terminato la prima fase). Se penso a quanti piccoli campi di calcio ci sono nei nostri piccoli Comuni per sostenere un sano sport dilettantistico rivolto specialmente ai giovani come sana attività e protezione da pericolose devianze che ben conosciamo, allora penso che sarebbe giusto eticamente, e possiamo dire anche sportivamente, che quanto incassato sarebbe anche da dire quanto perso - vada proprio a questa sana attività dilettantistica ed alle associazioni che tanto si impegnano e che tanto sono state ingannate, e poi disilluse, dalla Nazionale.

È stata una *full immersion* di confronto con le associazioni che rappresentano i vari settori del Paese e di confronto tra maggioranza ed opposizione, entrambi seri e costruttivi. Abbiamo lavorato senza limitazioni, e per questo vorrei fare un plauso al relatore e presidente della Commissione, che ha consentito indistintamente a tutti di dare un apporto.

Concludo con una riflessione sulle famiglie. C'è una stretta delle famiglie sui consumi: il clima di *austerity* colpisce, ad esempio, tempo libero e cultura; si salva solo l'abitazione. Cala la spesa alimentare, specialmente al Sud, mentre la spesa non alimentare risulta fortunatamente

colleghi, ci troviamo di fronte ad un voto di fiducia che ancora una volta mette a nudo la fragilità del Governo Berlusconi sia al suo interno, ormai divorato dalle divisioni, dalle inchieste, dai comitati d'affari e dalla ricerca ossessiva delle leggi *ad personam*, sia nel rapporto parlamentare con l'opposizione, vista come un fastidio piuttosto che come realtà con cui confrontarsi per il bene comune a colpi di progetti e proposte, sia, ancora, nei confronti della società italiana, ormai incredula, sfiduciata e portata agli estremi con un conflitto senza precedenti, ad esempio con i presidenti delle Regioni. Si tratta di tre limiti pesanti per un Governo formato da una larga maggioranza, ormai priva di coesione e reale capacità di governare una fase delicatissima della crisi economica del nostro Paese. Dopo due anni di ostinato negazionismo, vi siete svegliati, o meglio, siete stati costretti a svegliarvi dall'energico richiamo, formulato formalmente dagli organismi comunitari, sostanzialmente dalle scelte della Merkel, e siete corsi a mettere su una manovra contraddittoria: debole sui punti strutturali della spesa pubblica italiana e feroce con i disabili, con i giovani, con l'Abruzzo, con le forze dell'ordine, con il Mezzogiorno virtuoso, con il sistema intero delle autonomie locali. Attenzione: nella società italiana, anche nella parte più debole, è ben presente la consapevolezza della necessità di una manovra finanziaria in grado di reagire al debito pubblico che con le vostre scelte avete posto fuori controllo, tenuto conto dell'evolversi insidioso del ciclo della crisi internazionale che colpisce in particolare i Paesi europei e, tra essi, i Paesi più deboli, ad alto debito pubblico. In sostanza, è il come stare nella crisi e il come uscirne che non convincono. Non avete una grande idea, non avete una rotta, non avete una visione strategica per accompagnare e guidare il Paese fuori dai suoi limiti strutturali e dalle difficoltà in cui si trova, anche per la dinamica internazionale. Nella crisi ci si può stare in due modi. Il primo è un approccio classico, tipico dell'andazzo che ha avuto l'Italia negli ultimi decenni, tranne in alcuni brevi periodi: reagire tamponando, mettendo pezze, provando a limitare i danni; alla spesa corrente elevata ci si limita a rispondere tagliando, non riformando radicalmente la spesa pubblica e lo Stato.

un sistema di tagli che ormai raschiano il barile e non incidono sui problemi di fondo della formazione del debito dell'inefficienza del sistema e sulle capacità competitive e di crescita del nostro sistema produttivo e dei servizi pubblici. Anzi, anche al vostro interno non sono mancate voci autorevoli che denunciano addirittura la crescita della spesa corrente, la diminuzione radicale degli investimenti pubblici e la stessa crescita delle entrate. Insomma, Italietta eravamo prima della crisi, Italietta siamo dentro la crisi e, ancora peggio, Italietta rischiamo di essere dopo la crisi, qualora dovessimo uscirne, con tassi di crescita bassissimi, alto debito pubblico, spesa pubblica inefficiente, elevata divisione territoriale, scarsa coesione sociale, abbandono dei giovani e delle donne. È necessario un altro approccio alla crisi. Bisogna sposare l'idea che la crisi deve trasformarsi in una risorsa per riformare radicalmente il Paese, liberandolo dai suoi vecchi vizi e liberando tutte le sue stupende qualità e potenzialità. alcuni esempi di due diversi approcci alla crisi. L'Italietta dei tagli delle risorse alla sicurezza fa mancare anche a questo settore i beni più essenziali, ad esempio gli straordinari, la benzina per le automobili di servizio, un numero adeguato di pattuglie nel controllo del territorio. L'Italia delle riforme radicali riorganizza invece le innumerevoli forze di polizia, ma ancor di più ne riduce il gran numero complessivo, evitando ridicole sovrapposizioni e un numero di dirigenti e generali per forze di polizia da operetta. altro esempio: l'Italietta dei tagli lineari riduce il servizio giustizia, tanto che mancano 1.250 magistrati previsti dagli organici.

Poi il Ministro della giustizia viene in Commissione bilancio e ci propone la via dei precari, chiamati ausiliari, per smaltire l'arretrato in sede civile. L'Italia delle riforme fa altre scelte, più moderne, che migliorano il servizio giustizia e fanno ridurre la spesa pubblica. Mi riferisco alla necessità di rivedere radicalmente i tre gradi di giudizio.

un altro esempio: l'Italietta degli sprechi lo annuncia, ma non ha il coraggio di abolire le Province e lascia in piedi enti e meccanismi di intermediazione della politica. volte, di intermediazione burocratica e clientelare, e in molti casi anche affaristico-mafiosa. L'Italia delle riforme abolisce le Province, valorizza i territori,

del governo assistenziale della spesa pubblica e dell'intermediazione perversa di tipo burocratico, clientelare e - ripeto - spesso affaristico-mafioso. Questa Italietta non c'è più: l'Italia duale è dannosa sia per il Nord che per il Sud. poco vale, come spesso e a ragione si fa nel mio Sud, declinare i torti subiti, spiegare e dettagliare bene i falsi investimenti che sono stati fatti. Non serve fare questo lavoro, ma occorre denunciare la causa, andando a monte e spiegando che l'Italia duale è un danno per tutto il sistema Italia. Naturalmente lo è di più per il Mezzogiorno, che ha subito questo approccio così perverso sul piano strutturale, ma è un limite per tutti, che va superato. Ecco perché dobbiamo imboccare un'altra idea, idea, più matura e più forte. Dobbiamo avere il coraggio di ridefinire il patto che tiene insieme l'Italia. Ci vuole un'altra unità d'Italia, tutte le Regioni debbono diventare terra di produzione, in cui il Mezzogiorno non deve essere illuso, come è stato fatto anche in questa manovra, con delle scelte che in apparenza pensano al Mezzogiorno, ma che in sostanza provano a prenderlo in giro.

Presidente, nel nostro Paese c'è sì la consapevolezza che una scelta severa, rigorosa, dolorosa va fatta, ma non si vuole essere presi in giro. Si vuole un altro Governo. Si vuole un altro approccio. È quello che dobbiamo costruire.

due anni di Governo Berlusconi, è chiaro che c'è un problema strutturale, e noi dobbiamo mettere davvero mano, nel profondo, all'indebitamento del nostro Paese.

le Regioni, le Province, i Comuni, gli uffici periferici dello Stato, le camere di commercio. Non ci facciamo mancare nulla! E pensiamo che dopo aver accumulato un debito di questo tipo ne veniamo fuori con questa manovra? Non sarà così: purtroppo non sarà così. Non voglio fare il profeta di facile sventura e nemmeno sottopormi al ridicolo, però non sarà così. Lo sappiamo tutti che non sarà così.

Noi proponiamo le cose che abbiamo detto per l'immediato, che sarebbero più efficaci. Al tempo stesso vi proponiamo di mettere mano in maniera seria all'organizzazione di questo Stato. Quella è la vera sburocratizzazione. Altro che articolo 41! Le Province, le prefetture, le camere di commercio devono continuare ad esistere? Questo è un Paese in cui le riforme hanno sempre aggiunto. Per forza che oggi la spesa pubblica non la controlla più nessuno! Dobbiamo cominciare a togliere qualcosa.

Perché non si cerca di dialogare e di avere un confronto serio. Questo è il momento. Di fronte a questa crisi e a tutti problemi che abbiamo non c'è mai stato uno scontro così duro tra maggioranza e opposizione, e all'interno della maggioranza e anche all'interno dell'opposizione. Noi di fronte a questa situazione invece avremmo bisogno di ricucire, di ricomporre e di affrontare questioni davvero strutturali di questo Paese. Vengo all'evasione

Abbiamo il federalismo fiscale. Mettiamo mano davvero ad una riforma seria del fisco. Diceva il collega Giaretta che sono troppo pochi a pagare troppo. cento degli italiani possiede il 40 per cento della ricchezza. Bisogna andare ad una redistribuzione della ricchezza in questo Paese. E lo si fa attraverso una grande riforma fiscale che dia anche un senso civico. Guardate,

altre. Guardiamoci in faccia e dialoghiamo in maniera diversa: abbiamo opinioni diverse, ma di fronte a una crisi come questa bisogna sicuramente avere un confronto e una dialettica diversi, perché molto probabilmente così possiamo fare l'interesse del nostro Paese nella maniera migliore.

Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo c'è stata, nella vicenda che sta ingloriosamente per concludersi, un'evidente confusione tecnica che però stavolta ha superato i limiti della decenza. In una manovra già nata male, perché iniqua nella distribuzione dei tagli di spesa e incerta nella quantificazione delle voci di entrata, si sono mano a mano moltiplicati gli emendamenti sulle materie più astruse e disparate. A colpi di "refuso" quotidiano e di *blitz* notturni di fugaci *peones* e audaci relatori si sono aggiunte e sottratte impreviste stangate sulle assicurazioni e improbabili riforme del processo civile, intollerabili batoste sulle tredicesime e incredibili abbattimenti degli stipendi RAI. Nessuno ha mai negato che stiamo attraversando una crisi di portata globale come non si era mai vista o, per lo meno, nessuno dai banchi dell'opposizione, visto che dai banchi della maggioranza per mesi si è continuato a dire che andava tutto bene. Oggi, finalmente, ci si accorge che bisogna correre ai ripari e qual è la vostra risposta? Una manovra pesante che colpisce duramente categorie già ampiamente gravate da sacrifici: i giovani, innanzitutto; i lavoratori della pubblica amministrazione (una categoria sulle cui spalle alcuni Ministri hanno costruito addirittura la propria immagine) in particolare delle forze di polizia e dell'istruzione; tutta quella grande fascia di popolazione a cui Regioni e Comuni non potranno più offrire i servizi normalmente erogati. Tutti i richiami al buon senso, anche da parte di sparuti esponenti della maggioranza e dai Presidenti delle Regioni governate dal centrodestra, sono purtroppo caduti nel vuoto. E, ancora una volta, sottoponete il Parlamento al degradante stratagemma del maxiemendamento e della fiducia. È l'ennesima presa in giro dell'istituzione parlamentare da parte del Governo! Ieri abbiamo parlato della vergognosa vicenda dei disabili, oggi ne raccontiamo un'altra. Il canovaccio è lo stesso, ma questa volta i protagonisti erano addirittura i bambini. La manovra già taglia di fatto gli insegnanti di sostegno. Per rendere il tutto addirittura migliore (si fa per dire) era stato approvato dalla Commissione un emendamento firmato dai senatori Esposito e Latronico che prevedeva l'aumento del numero massimo di bambini nelle classi frequentate da alunni con disabilità. Il limite massimo (lo ricordiamo), per ovvi motivi di gestione della classe da parte degli insegnanti, è di 20 alunni. Con l'approvazione dell'emendamento in questione la prospettiva era quella di classi sempre più sovraffollate in cui la qualità dell'istruzione e dell'inclusione scolastica sarebbero state fortemente ridotte. Un atto, quindi, gravissimo che andava a colpire, ancora una volta, i più deboli. Un danno che avrebbe riguardato non solo gli alunni disabili (come se già questo non bastasse!) ma tutti i bambini e che avrebbe provocato un numero altissimo di contenziosi, ineluttabilmente persi dalle amministrazioni scolastiche e, dunque, un aggravio perfino per le finanze pubbliche. Altro che risparmi! In risposta alle ovvie proteste delle associazioni, ieri in serata è arrivata l'impacciata marcia indietro dei due presentatori che in una nota precisano: «Lo scopo e l'obiettivo è quello di ridurre il numero degli iscritti all'interno delle classi in cui ci sono alunni affetti da disabilità. Perciò non c'è volontà di penalizzare i disabili nelle scuole, piuttosto quello di favorire l'apprendimento e la scolarizzazione di questi grazie a classi sempre meno affollate». Peccato che l'emendamento esprimesse l'esatto contrario! Per fortuna anche in questo caso la norma è stata eliminata. Ma la domanda è sempre la stessa: è possibile che per raggranellare risparmi risibili si vadano a colpire anche i i minori, per giunta disabili? È ammissibile una tale cialtroneria e un tale pressappochismo sui temi sociali? Sulle pensioni, abbiamo assistito ad un altro balletto con la ben nota vicenda del cosiddetto refuso. Ieri il Ministro dell'economia si è premurato di far sapere quello che già tutti avevano capito: la storia del refuso era l'ennesima commedia per nascondere una decisione impopolare di cui nessuno, a cominciare evidentemente dal Ministro del lavoro, voleva assumersi la responsabilità. In alternativa dovremmo concludere che il Ministro dell'economia agisce senza nemmeno avvisare il proprio collega Ministro del lavoro. Quest'ultimo peraltro non sembra aver prestato molta attenzione ad una serie di temi a nostro avviso legati necessariamente alla scelta, che noi tuttavia ribadiamo come necessaria, dell'innalzamento dell'età pensionabile delle donne. Con i nostri emendamenti chiedevamo, ad esempio, un'attenzione particolare al tema delle disparità in ambito lavorativo di cui sono vittime le donne e alle dinamiche di cura dei bambini e degli anziani che gravano in gran parte sulle stesse. Riteniamo che sia necessaria una seria riflessione sulla conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro e l'adozione di misure concrete in tal senso. Se da un lato l'Italia è chiamata a raggiungere l'obiettivo della parificazione dell'età pensionistica tra uomini e donne, dall'altro non sono indifferenti, anzi sono indispensabili, misure di riforma del *welfare* e della previdenza in grado di eliminare contestualmente le condizioni che sono all'origine della differenza di età pensionabile, dissipando il rischio di aggiungere ingiustizia a disuguaglianza. È noto che in Italia le donne svolgono molto lavoro non pagato, a fronte di una vita lavorativa remunerata più corta, che ha come conseguenza una ricchezza pensionistica più ridotta. È indispensabile prendere atto che quelle di loro che si fanno carico di responsabilità familiari, di cura e della maternità, hanno una vita lavorativa complessivamente più lunga e pesante di quella degli uomini, con periodi di concentrazione spesso insostenibili e per cui pagano prezzi economici e professionali elevati. Sarebbe dunque necessario destinare a misure sia di sostituzione (tramite i servizi) che di riconoscimento del lavoro di cura (tramite congedi remunerati e contributi figurativi) i risparmi ottenuti con l'innalzamento dell'età pensionabile delle donne. Ciò consentirebbe anche di non distinguere genericamente tra donne e uomini, ma tra chi - donna o uomo - si prende cura dei figli o svolge attività di cura per persone non autosufficienti per età o malattia e chi no. L'Italia è in Europa tra i Paesi con i risultati peggiori in termini di differenziali di genere, in particolare con riferimento a lavoro e politica; l'occupazione femminile è molto lontana dagli obiettivi di Lisbona. Questo evidenzia, specialmente per il nostro Paese, un potenziale di crescita che un maggiore e migliore impiego delle capacità femminili consentirebbe di mettere a frutto. Chiudere il *gap* tra presenza maschile e femminile nel mondo del lavoro contribuirebbe anche ad alleviare il problema pressante della sostenibilità delle pensioni: l'aumento del numero degli occupati fra le persone in età lavorativa, infatti, ridurrebbe il cosiddetto «rapporto di dipendenza», ossia quello fra pensionati e lavoratori. Vanno ridotte ed eliminate le condizioni che producono il *gap* reddituale e contributivo tra donne e uomini, eliminando le discriminazioni di genere che ancora esistono nel mercato del lavoro ad ogni livello, dall'accesso alle forme contrattuali alle possibilità di carriera, rafforzando le politiche di conciliazione, per donne e uomini, dai servizi di cura per la prima infanzia e per le persone non autosuffìcienti ai tempi scolastici, che tengano conto del fatto che oramai nella maggioranza delle famiglie entrambi i genitori - o l'unico genitore presente - sono occupati. L'Italia, al contrario, è molto lontana dall'obiettivo europeo per il 2010: almeno 33 posti nei nidi pubblici ogni 100 bambini. Il nostro Paese, infatti, si ferma all'11,4 per cento, contro il 25-30 per cento del resto dell'Unione Europea. Per quanto riguarda l'aspetto più direttamente legato all'età pensionabile, una contestuale riforma del *welfare* deve contenere il riconoscimento di un adeguato valore economico al lavoro di cura e alla maternità, soprattutto sotto forma di contributi figurativi, come ho già detto, sulla scia di altri Paesi europei. Sono questi gli interventi a cui avevamo chiesto di destinare le maggiori risorse derivanti dalla implementazione dei provvedimenti di parificazione dell'età pensionistica per uomini e donne nel pubblico impiego. Mi rendo conto che forse queste sono argomentazioni eccessivamente tecniche in questo momento, ma credo siano necessarie per marcare, ancora una volta, la distanza tra chi fa proposte concrete e aperte nel merito dei problemi e chi si affida ai trucchetti dei «refusi»

c'è un convitato di pietra a cui dedicherò i minuti del mio intervento: il ministro Tremonti, il vero *dominus* della politica e delle scelte più significative di questo Governo, che ha voluto segnare con la sua filosofia anche questa manovra finanziaria, non ascoltando non solo le proteste, numerose e motivate, ma nemmeno alcuno dei contributi di merito che si sono levati in queste settimane in tutto il Paese, a cominciare dall'opposizione parlamentare, che ha voluto confrontarsi avanzando proposte che, a saldi invariati - come si è spesso detto in questi giorni - potessero rendere la manovra più equa, e soprattutto più utile al futuro del Paese. Ma il *dominus* non ne ha voluto sapere e questa manovra rinuncia alla sfida principale che il Paese ha dinnanzi, e che è rappresentata dalla necessità di riprendere la strada della crescita dopo anni di difficoltà e di stagnazione, culminati nella recessione degli ultimi mesi. Nessuna prospettiva di crescita del Paese, però, può prescindere dalla riproposizione di una questione che il Governo Berlusconi-Tremonti ha, con lucida caparbietà, inteso cancellare dal proprio orizzonte programmatico e, direi, finanche culturale: il Mezzogiorno del Paese. Proprio il ministro Tremonti ha raggiunto l'apice di questo suo atteggiamento, culturale prima ancora che politico, nei giorni scorsi, tradendo la sua vena di autentico antimeridionale, scadendo dalla sua abituale saccenza alla volgarità, dando del cialtrone a chi dal Mezzogiorno si permette di contestare le sue scelte. Da molti anni, ormai, dall'interno dello stesso Mezzogiorno si sono levate così tante voci critiche sui limiti delle classi dirigenti locali nell'utilizzo delle risorse pubbliche, spesso disperse in mille rivoli e talvolta terreno di corruttela e di malaffare, che davvero appaiono irricevibili e fuori dal tempo tali lezioni, che solo una memoria corta può rendere in qualche modo credibili. Peraltro, tale lezione arriva da chi ha operato con precisione chirurgica, in soli due anni, una colossale distrazione di risorse pubbliche nell'ambito dei cosiddetti fondi FAS (circa 28 miliardi) che per l'85 per cento erano destinati al Mezzogiorno, verso altri scopi, come ripetutamente abbiamo richiamato anche in quest'Aula. D'altro canto, è stata alimentata in questi anni una spesa corrente spesso volta a tutelare le clientele e il consenso elettorale della maggioranza di Governo: dalle multe dell'Unione europea agli allevatori padani sulle quote latte, che tornano in maniera anche ignominiosa in questa ennesima manovra finanziaria, alla copertura dei buchi di bilancio del Comune di Catania; dalla copertura dell'eliminazione generalizzata dell'ICI sulla prima casa alla vicenda Alitalia. E poi questa maggioranza e questo Governo sono stati quelli che, animati da una sorta di logica punitiva, bloccato i piani attuativi regionali dei fondi FAS, circa 18 miliardi di euro, che, pur avendo superato l'istruttoria tecnica del Ministero dello sviluppo economico, non sono ancora arrivati al CIPE, se si esclude quello della Sicilia, approvato lo scorso anno, nel pieno di una *bagarre* tutta interna al PdL. E poi, ancora, è stato svuotato il credito d'imposta, strumento moderno ed efficace di sostegno agli investimenti se svincolato da procedure e da mediazioni amministrative, ripristinando la vecchia e fallimentare logica discrezionale e i pesanti adempimenti amministrativi del passato, a danno del sistema di imprese meridionale. Insomma, direi al ministro Tremonti, se fosse qui, sostanzialmente smantellato un intero ciclo di programmazione (2007-2013) condiviso negli anni passati tra Regioni e Stato nazionale, sostituendo a tutto ciò la politica dell'annuncio, una politica sostanzialmente vuota e inconsistente. Che fine ha fatto infatti l'epocale Piano per il Sud annunciato la scorsa estate e che doveva essere presentato lo scorso dicembre sotto la responsabilità del ministro Scajola? E che fine ha fatto la Banca del Sud, una delle perle della fertile fantasia del ministro Tremonti? Piuttosto spieghi, il nostro, da presunto campione dell'efficienza e della qualità della spesa pubblica, come mai in questi due anni è aumentata di 20 miliardi la spesa pubblica, e come mai in questi ultimi anni i trasferimenti ordinari ripeto, dallo Stato alle Regioni meridionali sono scesi sotto l'ultimo Governo Berlusconi addirittura al 35 per cento. Una percentuale ben al di sotto di quel 45 in sede di programmazione nazionale negli anni passati: un vincolo, peraltro, di cui questo Governo ha pensato bene di liberarsi appena insediatosi due anni fa! C'è in tutti questi dati una verità storica che negli anni si è andata consolidando, e che Tremonti ed una diffusa letteratura cercano di nascondere: di fronte al continuo sottodimensionamento dei trasferimenti ordinari, i fondi comunitari hanno progressivamente perduto l'effetto di "addizionalità", assumendo sempre di più le caratteristiche di vera e propria finanza sostitutiva, che ha di fatto compensato il *deficit* di spesa ordinaria. C'è in tutto questo non solo l'opera ragioneristica di chi intende far quadrare i conti dello Stato di fronte ad una grave crisi finanziaria, trascurando le ragioni storiche di una parte del Paese ed una crescente questione sociale fatta di crisi produttive, perdita di posti di lavoro, calo dei consumi, disagio giovanile. C'è dell'altro: ovvero l'idea che, in nome di errori, presunti o accertati, che nei decenni sono stati compiuti nel dare risposte a volte sbagliate o inadeguate, si possa definitivamente eliminare dall'agenda del Governo nazionale del Paese una questione, quella meridionale, che è ancora, a nostro parere, una grande questione nazionale, la più grande. Questa manovra, per il notevole impatto finanziario, per essere la risposta italiana ad una crisi che coinvolge l'intera Europa, doveva sì rappresentare l'occasione per mettere in ordine i conti, ma allo stesso tempo poteva riavviare un processo di crescita che, tra le altre cose, valorizzasse pienamente le potenzialità del Mezzogiorno. In questa direzione andavano le nostre proposte: dal progressivo reintegro dei Fondi FAS ai crediti d'imposta, dal potenziamento delle infrastrutture portuali e ferroviarie alla ricerca, dal sostegno al credito per le piccole e medie imprese all'occupazione giovanile, all'allentamento del Patto di stabilità per favorire il rilancio della spesa in conto capitale di enti locali e Regioni. Invece avete scelto di volare basso, troppo basso: le zone a burocrazia zero, uno strumento inutile; il taglio dell'IRAP, una presa in giro. Di fronte a tutto ciò, il combinato disposto - dovete saperlo del taglio dei trasferimenti ordinari al Mezzogiorno con i tagli feroci che sono stati operati in questi due anni ai fondi FAS porterà ad un grave dissesto...*(il

in confronto al Paese. In una parola, il dualismo nel nostro Paese si aggraverà anziché allentarsi. È questa una preoccupazione condivisa, o no? Ecco, questo avremmo voluto chiedere al ministro Tremonti, il convitato di pietra di questo nostro dibattito.

sottosegretario Giorgetti stamattina, in replica alla discussione generale, ha sintetizzato le differenze di impostazione tra le politiche economiche proposte con questa manovra dal Governo e quelle proposte nella relazione di minoranza dalle opposizioni. E le ha sintetizzate in modo molto semplice: il Governo il Governo cerca di affrontare i temi dello sviluppo abbassando le tasse; all'opposto, l'opposizione affronta le questioni aperte dai temi dello sviluppo proponendo l'aumento la pressione fiscale.

un'idea di fondo della politica economica che è abbastanza coerente e costante fin dal DPEF del 2008: è una politica economica che si propone di lasciare andare libere le energie dei mercati senza intervenire, teorizzando che i mercati

Se il tema fosse tagliare la spesa pubblica improduttiva e abbassare le tasse, penso che saremmo tutti d'accordo e potremmo concludere il nostro dibattito. In realtà, non è così. non abbassa le tasse: anzi, tendenzialmente - è utile dirlo anche a quelli che hanno applaudito la manovra - fino a tutto il 2013 le aumenta,

L'hanno detto tutti, e non voglio farla lunga su questo punto, ma i tagli lineari sono un premio alla spesa improduttiva e una punizione per chi è stato virtuoso e ha reso efficiente la macchina amministrativa. i tagli lineari colpiscono maggiormente le aree più virtuose del nostro Paese, quelle che sono state più formiche e meno cicale, quelle che hanno apportato più valore al reddito nazionale nel suo complesso.

imprese. Non basta per un'economia come la nostra, da molto tempo in crisi di produttività, delimitare il perimetro delle tasse. Esse sono solo una delle componenti delle politiche fiscali. Se poi nelle tasche delle imprese non rimane un euro per gli investimenti e si dice che si sono abbassate le tasse, quello che succede è che non si fanno investimenti, non si punta sul futuro e non si investe in tecnologia, in capitale umano e fisico. Il problema della nostra produttività risiede proprio nella necessità di far leva sulle tecnologie, sull'accumulazione di capitale, sul funzionamento dei mercati e delle istituzioni di governo dell'economia.

produttivi e produttori del prodotto interno lordo nel nostro Paese non può guardare a questa manovra se non con molto sconcerto. Dov'è finita la politica industriale? È un anacronismo della storia che appartiene alle politiche di programmazione degli anni Settanta e Dove sono le politiche industriali in un Paese che ha un così grave *deficit* di produttività? Per farla breve, credo sia necessario l'uso delle politiche fiscali, soprattutto nella loro funzione redistributiva.

ovviamente deve essere fatto dallo Stato, ma su alcune questioni si poteva e si doveva fare di più, e forse molto diversamente. Soffriamo di una inadeguata accumulazione di capitale fisico e umano; essa è andata di pari passo ad un redistribuzione del reddito a sfavore dei salari e dei profitti e a favore della remunerazione del capitale. La questione della tassazione con standard europei delle rendite e dei patrimoni più tasse, ma spostare le tasse dalla parte produttiva e che consuma di più verso le aree meno produttive e meno consumatrici. Così come le liberalizzazioni e il loro assetto regolatorio possono agire contro le rendite monopolistiche, pubbliche e private, ed ancora liberare risorse per gli investimenti

dentro la crisi internazionale, ma con una specificità assolutamente tipica all'interno di tale crisi. È un Paese che non cresce da molto tempo, e la manovra non affronta le questioni che sono da tempo aperte; anzi, talune vengono sollecitate in modo in modo anche populista e francamente un po' da presa in giro, come nel caso della semplificazione. Cosa c'entra la semplificazione con l'articolo 41 della Costituzione? Cosa c'entra il fatto che l'impresa sia sancita nella Costituzione e ne siano sanciti il ruolo e il compito sociale con la semplificazione normativa? Le semplificazioni si fanno molto più semplicemente, senza scomodare la Costituzione, basta volerle fare.

il Governo non aveva previsto, poi non ha compreso, poi non ha riconosciuto, continuando a muoversi come se l'Italia potesse stare al di fuori del contesto internazionale in cui si come se l'Italia non avesse i suoi problemi specifici, aggravati dal quel contesto internazionale. Non stavamo meglio degli altri: stavamo peggio, perché avevamo meno riserve positive da mettere a disposizione contro la crisi. Adesso vediamo che stiamo peggio, e questa manovra non basterà. *(Applausi

come altri colleghi del mio partito e dell'opposizione, preannuncio subito un voto nettamente contrario alla fiducia; non lo faccio in termini generali, perché alcuni alcuni interventi che mi hanno preceduto hanno già illustrato gli aspetti complessivi della questione, ma attiro l'attenzione solo su alcuni punti che considero importanti. In merito all'autocertificazione autodeterminata, che dovrebbe sostituire la DIA e che ha suscitato forte allarme, considero una vittoria dell'opposizione e dell'opinione pubblica il fatto che il Governo, nel testo definitivo, all'ultimo momento abbia fatto qualche passo indietro relativamente agli aspetti che sembravano più scandalosi o strambi. Mi riferisco, per esempio, alla possibilità delle università di rilasciare certificazioni in materia di

contrasto tra questa autocertificazione e la legislazione di salvaguardia del territorio in termini di piani paesistici, piani strutturali, regolamenti edilizi eccetera. C'è qualche miglioramento: sono stati portati a 60 i giorni per l'adozione dei provvedimenti; sono esclusi - grazie al cielo - dalla procedura semplificata tutti i casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici e culturali; i controlli *ex post* sono consentiti anche se il pericolo di danno non si configura come grave e irreparabile, come era scritto nel testo precedente. Consideriamo questo un ravvedimento operoso, però non è sufficiente a convincerci della bontà dell'impianto generale. C'è da dire che il modo di gestire territorio e paesaggio non può essere risolto con strumenti così eterogenei e sbrigativi e soprattutto poco conformi allo scopo. Temiamo anche che si sia trattato di un *ballon d'essai* per saggiare il grado di resistenza dell'opinione pubblica, che - grazie al cielo - si è fatta sentire: anche l'ANCE, le associazioni degli urbanisti e degli architetti hanno protestato. Ma i bisogni fondamentali di piani di tutela, di consolidamento e sostituzione del patrimonio edilizio non possono essere risolti nei termini che il provvedimento stabilisce su questo tema. secondo punto attiene alla questione del documento unico di regolarità contributiva. Si tratta di uno strumento importante ed efficace per contrastare il lavoro sommerso, che riguarda anche i lavori concernenti la manutenzione straordinaria, che prima erano soggetti alla DIA, titolo abilitativo edilizio. Questo documento unico di regolarità contributiva non deve essere sottoposto a *deregulation*, non può diventare uno uno strumento gravato da opacità. Uso questo termine perché spesso, nella manovra, i termini non sono chiarissimi e si può nutrire il dubbio che espressioni

deve essere inteso con riserva, perché dobbiamo aspettare a vedere se questa opacità della lettera della norma non serva poi a determinare scarsa chiarezza in sede di applicazione.

del decreto-legge e poi però nel testo depositato era scomparsa. Ora la vediamo riapparire nel maxiemendamento, nella stessa formulazione che era uscita dalla Commissione bilancio e sancita dall'emendamento del Governo. Non è chiarissimo perché ci sia stato questo andirivieni, questo metti e leva: cosa vorrà dire? dire? In sostanza per arrivare a una messa in sicurezza delle trattative che hanno per obiettivo la conclusione o la ridefinizione del debito o di un concordato preventivo rispetto ad azioni cautelari si aggiunge un intervento sui reati. Di fatto, si tratta di un allineamento del penale al civile. Questo mi risulta alquanto irrituale ed è causa di dubbi. Quale sarà il motivo? Il motivo buono potrebbe essere la volontà di mantenere in vita imprese in crisi, ma il motivo cattivo cela una domanda: a chi serve? Ci siamo abituati, in quest'Aula, ad esaminare provvedimenti dal destinatario incerto, espressioni poco chiare che poi celano il favore a qualcuno. Aspettiamo di vedere e di poter controllare che cosa succederà sulla base di queste formulazioni. In ogni caso, se si deve discutere di reati di natura fallimentare, perché non parlarne in Commissione giustizia?

del pagamento di Mondadori a CIR. È una questione annosa, fa parte delle tristezze della nostra vita politica. Il lodo Mondadori ha con sé una serie di conseguenze nebulose.

del contenzioso tributario relativo al lodo Mondadori. Ora - grazie al cielo - con questa ultima fuoriuscita dal testo ci viene risparmiato di sapere che il pagamento che Mondadori deve a CIR per lo scippo, l'esproprio proprietario esercitato da da Fininvest su Mondadori, non è più rinviato di sei mesi in sei mesi. Vedremo poi se la vicenda andrà a buon fine. Certo è che ogni aspetto, anche involontariamente, nell'esame di queste leggi e di questa manovra, anche se non volessimo ci fa tornare sempre, come di consueto,

che sostanzialmente questa manovra appare come una riduzione delle tasse per chi ha l'abitudine di non pagarle, mentre di fatto, come hanno già spiegato con grande competenza molti colleghi, le aumenta per chi già le paga e, nello stesso tempo, non crea risorse per lo sviluppo. Di straforo avete tolto l'ICI, una delle pochissime imposte di natura federalista; adesso scoprite che ne avete ancora bisogno, e nello stesso momento in cui dite che non mettete le mani nelle tasche degli italiani le

Avete continuato ad impoverire fin dall'inizio della prima finanziaria e senza rimedio la scuola, l'università e la ricerca. In questo modo fate venire a mancare la linfa fondamentale al nucleo essenziale che solo può garantire la ripresa dell'economia in questo Paese.

Ho chiesto di intervenire non tanto per ribadire alcune questioni che si riferiscono al carattere iniquo della manovra,

le colpisce in forma diretta come lavoratrici del pubblico impiego e come donne prossime alla pensione, e in maniera indiretta su tutte le questioni che hanno a che vedere con il *welfare*, soprattutto quello locale, e i servizi alla famiglia.

l'Expo con la candidatura di Milano, avrebbe dovuto inventarsi un qualche evento di portata nazionale per riuscire a fare una politica anticrisi. Questo Paese ha avuto la fortuna di avere in campo un progetto di questa natura e di averlo nell'area più importante, significativa e trainante: Milano e la Lombardia.

dovremmo consegnare le strutture pronte ai Paesi partecipanti nell'ottobre 2014, ma non è partito nulla.

Devono iniziare i lavori che interessano due linee di metropolitana e un prolungamento, due tratti di autostrada, un raccordo ferroviario per rendere accessibile l'area: mancano meno di quattro anni a questo appuntamento.

come si è visto per la Grecia e, volendo fare un confronto, come non si è visto per il Giappone o per altri Stati - dipendono dal debito del Paese, ma anche dalla sua credibilità internazionale. Allora, vorrei sapere se vogliamo mostrarci agli occhi del mondo come un Paese così in decadenza

siamo di fronte al fallimento del centrodestra che in quel territorio governa Regione, Comune e adesso anche Provincia ed è al Governo, ma non riesce ad uscire da questa situazione per una lotta di potere interna, legata solo alla spartizione degli affari.

*(PD)*. Signor Presidente, la crisi generalizzata della finanza pubblica nell'area occidentale richiede certamente azioni congiunte di entità rilevante. Possiamo affermare che una parte della manovra finanziaria sulla quale il Governo ha posto la questione di fiducia è stata scritta sotto dettatura dell'Unione europea. Se il rigore della manovra era inevitabile, oltre che auspicabile, non erano però inevitabili la dimensione e soprattutto i contenuti del provvedimento: fattori politici ascrivibili alle azioni (e alle mancate azioni) del Governo hanno peggiorato la situazione del Paese in cui la manovra si inserisce. Nei due anni di governo in questa legislatura si è nuovamente perso il controllo della spesa pubblica (quella spesa pubblica su cui questa manovra intende tardivamente intervenire) abbiamo assistito in particolare a un aggravamento del debito pubblico rispetto al prodotto interno lordo molto superiore all'effetto del calo del PIL. In due anni di questo Governo, le stime dimostrano che il livello dell'evasione fiscale è tornato a salire dopo la riduzione registrata nel precedente biennio di Governo del centrosinistra. bizzarre le scelte del Governo Berlusconi: ora, con l'acqua alla gola, si reintroducono misure di contrasto all'evasione che lo stesso Governo aveva cancellato; ora si torna a prevedere la tracciabilità dei pagamenti; ora si introducono e si valutano 7,5 miliardi di euro di nuove entrate, derivanti dalla lotta all'evasione (e di questa previsione, tra l'altro, è più che lecito dubitare). E prima? Prima, poiché la crisi secondo il Presidente del Consiglio non c'era (era ascrivibile a una percezione distorta della realtà, era di natura psicologica), l'evasione fiscale poteva essere tollerata, persino compresa, se non incoraggiata. Prima i capitali evasi e trasferiti all'estero potevano essere fatti rientrare a prezzi di favore (il 5 per cento, rispetto al 40 o al 50 per cento dovuto negli altri Paesi) e con garanzia di anonimato. poi le scelte del Governo che hanno ulteriormente peggiorato lo stato dei conti pubblici per dar seguito alle promesse elettorali del presidente Berlusconi: la completa eliminazione dell'ICI sulla prima casa per esempio, anche per i redditi e i patrimoni più elevati; il cosiddetto salvataggio dell'italianità di Alitalia, per esempio, che, sommando i debiti della compagnia che ricadono sullo Stato, i 400 milioni di euro di prestito non restituito e gli ammortizzatori sociali, è costato alle casse pubbliche ben più di 3 miliardi di euro. Potrei continuare. Adesso i nodi vengono al pettine; adesso non si può più far finta di niente; adesso si presenta una manovra pesante, manovra pesante, ma senza coraggio, senza la capacità di chiamare gli italiani a uno sforzo per uscirne migliori, per raggiungere insieme obbiettivi ambiziosi. Certo, per fare questo servirebbe un Governo capace di unire gli italiani, non specializzato nel dividerli. No, si chiamano i cittadini a sacrifici senza alcuna prospettiva, se non quella di restare a galla. Questa è una manovra dimessa, rinunciataria, che non cambia e che non riforma. Del resto, autorevoli Ministri di questo Governo - Tremonti, Sacconi e altri - in questi mesi hanno più volte teorizzato l'opportunità di non fare le riforme, mentre, al contrario, sarebbe necessario far leva sulla maggiore disponibilità al cambiamento, che esiste nelle situazioni straordinarie, per proporre vere politiche riformatrici. Per finire, vorrei fare un accenno al contenimento della spesa e ai tagli. Sarebbe ingeneroso non riconoscere che in questa manovra qualcosa (non molto) che va in questa direzione c'è. E noi dobbiamo sapere che senza una lotta decisa, feroce allo sperpero (che esiste) di denaro pubblico non si potranno, come invece si deve, ridurre le tasse e non ci sarà denaro per coloro che dello Stato hanno davvero bisogno. Anche un nuovo patto fiscale tra il cittadino e lo Stato non sarà possibile se molti cittadini pensano, in parte a ragione, che lo Stato butta dalla finestra o usa malamente una parte rilevante dei soldi delle tasse che chiede ai contribuenti. I tagli alle spese possono però essere veri o codardi, se mi passate il termine. Molti sono quelli veri che si potevano fare e non si sono fatti, soprattutto disboscando in modo selezionato la giungla di enti di cui si sono progressivamente riempite le varie articolazioni dello Stato, o eliminando quelle Province che coincidono (poco più) con le grandi città. Divertente il balletto sulle Province: prima si annuncia la soppressione di quelle più piccole, che sono quelle che spendono meno; poi si introducono criteri per salvarne alcune; poi quei criteri non bastano, perché il rischio di soppressione della Provincia di Bergamo fa venire l'orticaria al ministro Bossi; poi le Province da eliminare sono sei, poi cinque, poi tre; poi si demanda la decisione al nuovo codice delle autonomie; poi non se ne fa niente. Tagli veri dunque, mentre quelli codardi sono quelli di cui è invece piena questa manovra: tagli che consistono semplicemente nel mettere in altre mani la patata bollente. Tagli alle Regioni, che significano meno risorse per gli incentivi alle imprese, per il Fondo non autosufficienti, per le famiglie, per l'*handicap* e il sociale, per la casa, per il lavoro Tagli molto forti al trasporto pubblico locale, che significheranno per bus, metro e ferrovie locali aumento del costo dei biglietti o riduzione delle corse. Tagli ancora una volta ai Comuni, cioè ai mille servizi che i Comuni quotidianamente erogano e a quella parte del *welfare*, quello municipale, che più e meglio degli altri ha già saputo e dovuto autoriformarsi in questi ultimi 15 anni. E tagli E tagli all'ANAS, che si ripetono, ma si accompagnano all'assoggettamento al pedaggio dei raccordi autostradali gestiti dall'ANAS e all'aumento dei pedaggi sulle autostrade, con trasferimento all'ANAS dei relativi introiti, e al mantenimento della tassa sui passi carrai delle strade ANAS, spremendo malcapitati cittadini e piccole imprese. Anche per la natura di questi tagli operati dal Governo questa manovra finanziaria non ci piace.

Sottosegretario, «la fiducia è un atto di coraggio»: così il presidente Berlusconi annunciava a mezzo stampa l'ennesimo voto di fiducia. Altro che coraggio! In realtà questo ennesimo voto di fiducia nasconde una grande paura: nasconde il timore di confrontarsi con il Paese reale che in queste ultime settimane ha assediato i palazzi della politica chiedendo un confronto serio con il Governo sulle gravi misure previste dalla manovra, misure che avranno una dura ricaduta sulle condizioni di vita reali di tanti cittadini italiani ed in particolare dei cittadini più deboli: i cassintegrati, i pensionati, i precari, i disoccupati. Misure che, come diceva prima il collega Sangalli, sono devastanti per la piccolissima impresa, soprattutto per quella mononucleare. La fiducia come atto di codardia: una porta sbattuta in faccia a (chiamiamoli con i loro nomi) insegnanti, medici, poliziotti, ricercatori, maestre che invano in questi giorni hanno cercato un dialogo capace di scongiurare misure che determineranno nel nostro Paese meno sicurezza, meno competitività, meno sviluppo, minori servizi sociali per i cittadini. Una porta sbattuta in faccia ai Presidenti delle Regioni, che inutilmente, anch'essi, ma responsabilmente ed in maniera unitaria hanno tentato di spiegarvi, conti alla mano, che i tagli previsti dalla manovra si tradurranno in duri tagli ai livelli di assistenza, alla sanità pubblica, al trasporto pubblico locale. Una fiducia, quella che siamo chiamati a votare, che segna anche un duro colpo alle relazioni istituzionali nel nostro Paese e allo stesso progetto federalista. Ma con questa ennesima fiducia il Governo si assume in pieno anche la responsabilità politica di chiudere ogni possibile dialogo con l'opposizione.

Si tenta, evitando la discussione e il confronto, di nascondere all'opinione pubblica che a fine anno, grazie alle misure introdotte dalla manovra, decine di migliaia di lavoratori precari della pubblica che stanno esaurendosi le risorse per gli oltre 600.000 cassaintegrati e che nella manovra non c'è nulla per gli ammortizzatori sociali; che la disoccupazione, in particolare quella giovanile, continua a crescere e nella manovra non c'è nulla per il sostegno alle imprese e all'economia; che si umiliano ancora una volta i dipendenti pubblici (insegnanti, medici, infermieri, poliziotti) con un taglio secco, l'ennesimo, alle loro retribuzioni. Un taglio orizzontale, che non terrà conto della produttività e dell'efficienza nella pubblica amministrazione, che ne colpirà soprattutto quella parte che funziona, alla faccia della tanto osannata riforma della pubblica amministrazione voluta dal ministro Brunetta, che in questi mesi mi pare scomparso.

politici ministeriali; un progressivo accorpamento degli uffici periferici dello Stato; una riduzione di spesa per la Presidenza del Consiglio dei ministri e della Protezione civile, con particolare riguardo alla moltiplicazione dei posti negli organici dirigenziali, al contenimento dei *budget* per le strutture di missione per un importo non inferiore a 10 milioni di euro, alla riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari;

Ma a fronte di proposte concrete, di cui non potremo discutere a causa del voto di fiducia, abbiamo dovuto assistere ad un balletto insopportabile proposto dai Ministri di questo Governo. Refusi su argomenti decisivi per la vita di tanti lavoratori, come quello sui 40 anni di contributi per accedere alla pensione. Ieri il ministro Tremonti ha detto che non era un refuso: ci ha provato, aveva fatto il gioco delle tre carte. È questo il modo di essere seri verso lavoratrici e lavoratori che per 40 anni hanno lavorato in posti disagiati, dove la salute spesso è messa in discussione? Stiamo parlando del lavoro dipendente privato di operaie e operai, in particolare dei settori tessile e meccanico.

pelle e che, concluso lo *show* mediatico sotto i colpi degli scandali, per veder riconosciuti i loro più elementari diritti sono stati costretti a urlare per far sentire la loro voce. Non hanno fatto così furbetti che, a differenza della stragrande maggioranza dei loro colleghi, ancora si ostinano a non voler pagare le multe sullo sforamento delle quote latte. È una vergogna! Lo abbiamo detto più volte. Eravamo disponibili, data la situazione nazionale ed internazionale, a fare la nostra parte. Ci avete risposto di no, come avete risposto di no alle Regioni, ai sindacati, alle forze sociali. Vi siete assunti e vi assumete una grave responsabilità. Vi nascondete dietro il voto di fiducia, ma non potete più nascondere il crescente disagio che c'è

sulla quale domani voteremo l'ennesima fiducia (la 34a in 26 mesi, dunque una media di 1,3 fiducie al mese), non affronta alcuno dei problemi gravi di un Paese stremato, che non vede alcun bagliore oltre il tunnel della crisi; anzi conferma i tagli biennali già previsti dal decreto-legge del Governo a carico delle Regioni (pari a 4 miliardi per il 2011), dei Comuni e degli enti locali. Vi siete sempre vantati di non voler mettere le mani nelle tasche degli italiani, ma da quando vi siete insediati vi avete messo anche i piedi, favorendo caste, cricche, evasori, riciclatori, speculatori, affaristi, faccendieri e tutti coloro che praticano l'omertà più assoluta. La situazione della finanza pubblica non è delle più rosee: la pressione fiscale continua ad aumentare in coincidenza con la diminuzione del PIL; continua inarrestabile la corsa del debito pubblico, che sfonda quota 1.827 miliardi di euro, crescendo di circa 15 miliardi rispetto ai 1.812 miliardi di aprile e raggiungendo i 30.451 euro a carico di ognuno dei 60 milioni di cittadini o, se si preferisce, di ben 83.050 euro per ognuna delle famiglie italiane. Il debito è cresciuto di 65,875 miliardi di euro dal dicembre 2009: in soli 5 mesi è aumentato del 3,7 per cento ad una media di 13,2 miliardi di euro al mese, nonostante tassi di interesse tra i più bassi Voglio ricordare che se non si arresta questa deriva, a fine anno il debito può toccare 2.000 miliardi di euro. E' da tempo che si chiede un'incisiva azione per ridurre il debito, soprattutto seguendo politiche di tagli a sperperi, sprechi e finanziamenti a fondo perduto, che nel 2009 si sono attestati a ben 39 miliardi di euro; però non si fa nulla. L'enorme massa di debito pubblico potrebbe ridursi utilizzando le dismissioni di oro e le riserve della Banca d'Italia, come hanno fatto finora tutti i Paesi dell'area euro, se il capo di tutti gli oligarchi, quel governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, (che qualche sera fa ha partecipato alla famosa cena con il cardinal Bertone ed il capo delle Assicurazioni Generali nell'ampio attico di Propaganda Fide nei pressi di piazza di Spagna) profittando del rialzo dell'oro, vendesse, in base anche ad alcuni accordi, riserve per ben 104,134 miliardi. Questa è una manovra che non tocca i capitalisti delle bollette e dei pedaggi e quei predoni coraggiosi,

E mentre il presidente Obama, la Merkel e Sarkozy e perfino il Governo conservatore inglese cercano di far pagare i costi della crisi anche ai banchieri che l'hanno provocata, il Ministro dell'economia non sfiora neppure i nostrani *bankster*, che anzi sono stati premiati con la nomina di un uomo del presidente Bazoli alla Cassa depositi e prestiti. Far pagare i banchieri ed un sistema bancario tra i più vessatori, fraudolenti ed inefficienti del continente, che ha resuscitato il pizzo della commissione di massimo scoperto, è un tabù invalicabile per il Governo e per il Ministro dell'economia. Voglio ricordare che negli ultimi cinque anni, su un totale di 6.155 miliardi di euro di finanziamenti per cassa, la commissione di massimo scoperto, arbitrariamente conteggiata dal sistema bancario ai debitori al di fuori dei tassi soglia regolati dal comma 4 dell'articolo 644 del codice penale, ammonta a 181,9 miliardi di euro. E secondo le rielaborazioni su dati Bankitalia, tra il 2005 e il 2009 il sistema bancario ha beneficiato annualmente di oltre 35 miliardi di euro a titolo di commissioni di massimo scoperto. Per non parlare dei *credit default swap* (CDS), che a fine 2009 erano cresciuti del 2,3

I giochetti e le scommesse dei banchieri nostrani, analoghi a quelli effettuati dagli altri banchieri amanti del gioco d'azzardo che acquistano i CDS, contratti con cui ci si assicura dal rischio fallimento di un'emittente di titoli, contribuiscono a portare alla rovina l'economia reale ed a picco la stabilità dell'euro; invece di arrestare questi giochetti da parte di banchieri che si comportano da biscazzieri, si continua in questo modo come se nulla fosse. Invece di far gravare i costi della manovra del tutto insufficienti per la gravità di una crisi occultata da almeno due anni - su lavoratori e pensionati, si poteva agire sui capitali "scudati" con una cedolare secca non si è fatto nulla. Si poteva introdurre un'aliquota dello 0,50 per cento sugli impieghi sterilizzati al 31 dicembre 2009, pari a 1.360 miliardi di euro, per ristabilire un minimo di equità nei pregressi rapporti contrattuali, in modo da generare un gettito di 6,8 miliardi di euro. Si poteva introdurre una tassa del 10 per cento sull'oro, come ritenuta di acconto sulle future dismissioni delle riserve auree, cosicché anche la cricca di banchieri e banche centrali, tra i principali responsabili della crisi, poteva concorrere al risanamento delle finanze pubbliche alleviando i costi che gravano sulle famiglie, per una cifra pari a 6,7 miliardi di euro.

Il Governo però non ha scelto questa strada. Questa manovra non sfiora neppure da lontano le consolidate oligarchie, i sepolcri imbiancati, le autorità cosiddette indipendenti con licenza di mercimonio, i grandi patrimoni, le grandi fortune, gli speculatori finanziari e quelle stesse banche che hanno prodotto una gravissima crisi, anche in Italia, facendo pagare a rate e con una specie di mutuo trentennale gli altissimi costi dei servizi bancari, tra i più elevati del mondo tassi sui mutui più alti dello 0,59 per cento rispetto alla media europea ed il credito al consumo con tassi maggiorati del 2,16 Non ci sono misure per i giovani e per quel popolo di precari che invecchia senza trovare speranze di lavoro, né banche che finanzino richieste di mutuo alle giovani coppie, che spesso vivono a carico dei veri e propri ammortizzatori sociali, che altro non sono che le famiglie le famiglie ed i risparmi dei vecchi. È una manovra iniqua, che non rilancia né lo sviluppo né il Sud bistrattato e dimenticato, né trova soluzioni definitive ai terremotati dell'Aquila - ricordo che c'eravamo quel giorno che sono stati picchiati dalla polizia, pur essendo manifestanti pacifici, cosa di cui bisognerebbe vergognarsi

di uno dei terremotati, ai quali una società di recupero crediti chiedeva di recuperare il credito per conto di Sky, i Non avete trovato soldi per le fasce più deboli, ai quali gli enti locali a secco dovranno tagliare i servizi sociali o inasprire le tasse, ma sono usciti dal cilindro del Ministero dell'economia soldi per i tanti furbetti del quartierino che hanno truffato lo Stato con le quote latte. Come tutti coloro che ritengono di essere autosufficienti

nell'elaborazione di proposte serie - 48,5 miliardi di euro - a carico di coloro che hanno prodotto la crisi, di coloro che non pagano mai il conto, per non far gravare i costi della crisi sempre sulla povera gente, su quelli che non ce la fanno. Per queste ragioni, e concludo signor Presidente, voteremo contro una manovra fatta di pedaggi, di tagli, che potrà anche avere l'approvazione dell'Ecofin, ma non ha il consenso della maggior parte del popolo degli italiani, di quei lavoratori e pensionati, di quei precari e disoccupati che continuano a soffrire i morsi di una crisi e a sopportare politiche economiche dissennate e molto spesso, come con lo scudo fiscale, criminali, addirittura immorali.

era la coniugazione del necessario rigore finanziario, che abbiamo sottolineato più volte, con l'equità sociale, tanto più dopo gli effetti molto gravi gravi di questa crisi, e con la ripresa della crescita della nostra economia. Serviva prima della crisi, tanto è vero che il Governo Prodi su questi binari aveva costruito la sua politica economica e di bilancio; serviva all'inizio della crisi, durante la crisi, e tanto più servirebbe oggi, stante la gravità della situazione economica nazionale ed internazionale che abbiamo di fronte. Ciò che serviva, inoltre, al nostro Paese era far coincidere, nei limiti del possibile, la riduzione della spesa, che ci deve essere, spesa che è continuata a crescere in questi due anni, con le riforme strutturali, come abbiamo detto in tutti i modi e in tutte le sedi e abbiamo ripetuto nel presentare e motivare le nostre proposte: rendere cioè la spesa pubblica maggiormente sostenibile, attraverso il, e contestualmente al, cambiamento della nostra pubblica amministrazione, molte volte pletorica ed inefficiente. Inoltre, occorreva ed occorre non smarrire mai un percorso di riduzione del debito, attraverso il meccanismo non soltanto nell'immediato di riduzione del deficit, ma di ricostituzione e poi di accumulo dell'avanzo primario. Anche in questo caso, un percorso che è stato interrotto, certo per effetto della crisi nel 2009, ma anche in virtù delle scelte che il Governo ha compiuto in questi anni. Si può dire che queste grandi esigenze del Paese e della finanza pubblica siano state soddisfatte con questa manovra? Penso di no. neanche i più accesi sostenitori di questa manovra direbbero ragionevolmente di sì, perché questa manovra produrrà una riduzione non permanente né strutturale della spesa corrente (e qui potremmo fare esempi molteplici), non produrrà uno snellimento a vantaggio dei cittadini e delle imprese della macchina pubblica, non produrrà un un impulso alla crescita della nostra economia; anzi, durante l'esame in Commissione, abbiamo accertato attraverso dati ufficiali che la manovra è depressiva, come è normale che sia

anni. Lo abbiamo detto in tutte le altre circostanze, a partire dalla manovra triennale che il Ministro dell'economia e il Governo vollero all'inizio di questa legislatura, e poi in occasione dell'esame e dell'approvazione di tutti provvedimenti durante questi due

Regole contabilistiche largamente condivise, una prassi consolidata nel tempo portava a ritenere che le nuove entrate derivanti dalla lotta all'evasione venissero portate a copertura dopo il loro effettivo e concreto conseguimento. Questa scelta, signor Presidente, rende da un punto di vista dell'attendibilità delle previsioni questa manovra assolutamente fragile poiché la componente a questo titolo indicata dalla manovra stessa non è affatto irrilevante. Ma abbiamo registrato - ed è questa l'altra novità - che le politiche che propone il Governo, certo difficili - per chiunque lo sarebbero state in questa fase fase storica - non sono più in sintonia con le aspettative del Paese, con ciò che servirebbe al Paese. Al contrario, abbiamo registrato vieppiù in questi giorni e settimane che le proposte ragionevoli, serie, argomentate, fondate e coperte che l'opposizione ha presentato, e di cui i colleghi che sono intervenuti prima di me hanno parlato, sono in sintonia con le necessità del Paese. del Paese. Tutti quanti noi ricordiamo come nel recente passato le posizioni che il Ministro dell'economia, pur da un punto di vista di politica di bilancio ed economica che noi non condividevamo, che veniva sintetizzata nella parola ripetuta più volte nelle Aule parlamentari, sembravano incrociare un'attenzione, un consenso, una qualche forma di sostegno da parte dell'opinione pubblica. Oggi non è più così, perché gli effetti della crisi si sono manifestati in tutta la loro gravità ed avevano bisogno di trovare risposte diverse: quelle che ci siamo sforzati di proporre proporre durante il lungo percorso, in Commissione e poi qui in Aula, di questa manovra. La riprova che così non è, cioè la riprova del fatto che le proposte del Governo, le politiche, le misure introdotte in questa manovra non incrociano più il consenso del nostro Paese

la possiamo ricavare dal fatto che lungo quattro settimane, 90 ore di lavoro serio ed approfondito che abbiamo fatto in Commissione, di fronte alle nostre precise e ragionevoli proposte, il Governo è rimasto silenzioso. È la prima volta, signor Presidente, che questo accade. Il Governo non ha argomenti per contrastare le ragioni che militano a sostegno della necessità di un'altra politica. L'altra novità, signor Presidente, è che con questa manovra sono ritornate le approssimazioni, la confusione, il tentativo - come veniva chiamato in gergo parlamentare - di assalto alla diligenza. Tutti ricordiamo il Ministro dell'economia che ci ha ripetuto più volte, da due anni a questa parte, «scordatevi le vecchie finanziarie». Che cos'è questa ? Che cosa è stata questa, con 1.200 emendamenti da parte della maggioranza? L'unica occasione nella quale il numero degli emendamenti da parte della maggioranza, quasi tutti di spesa, sono stati superiori a quelli proposti dall'opposizione. La maggioranza ha tentato di inserire di tutto; alla fine

capitoli di bilancio, tutte cose che il Presidente Azzollini ha cercato di arginare, ma alla fine si è dovuto arrendere alla pressione fortissima arrivata dalla maggioranza. Per fortuna, signor Presidente, l'opposizione e il nostro Gruppo hanno fatto un lavoro serio: hanno tentato di arginare il danno, e abbiamo ottenuto dei risultati e dei miglioramenti, che ci sono nella manovra: sono stati ricordati dai colleghi, e non voglio ritornare su di essi. Abbiamo evitato Mi riferisco, per esempio, a quella assurda riforma del processo civile che all'ultimo momento si voleva inserire nella manovra. Per fortuna, è stata espunta la riforma dell'autotrasporto che, al di là del merito, per il modo in cui era entrata era inaccettabile. È stata cambiata quella norma dagli effetti devastanti sulla riforma del procedimento amministrativo

tutti i procedimenti autorizzatori, compresi quelli su materie delicatissime quale la difesa nazionale, la sicurezza, la salute, l'ambiente, il paesaggio, i beni culturali e così via.

Noi abbiamo registrato passi avanti importanti in Commissione. Lo ha già fatto il presidente Marini oggi e lo faccio anch'io: ringraziamo il presidente Azzollini, i colleghi di maggioranza e il Governo per aver accettato quella ragionevole proposta di reintroduzione della zona franca urbana, con raddoppio delle risorse. Adesso la zona franca urbana può partire, non poteva perché non vi erano sufficienti risorse e strumenti. Si è fatto un passo avanti sulla rateizzazione delle imposte, ma c'è molto ancora da fare. Il tema della fiscalità va definitivamente sistemato, perché anche con questa formulazione il rimborso è insostenibile: da gennaio i cittadini e le imprese aquilane e del cratere dovrebbero pagare il corrente e rimborsare un decimo di di tutto il sospeso, il che non sarà sostenibile, e quindi occorrerà reintervenire prima della fine dell'anno. Soprattutto si è dimostrato che gli strumenti legislativi e finanziari

La ricostruzione non è partita; le risorse non sono immediatamente e ordinatamente disponibili; vi è incertezza su tutto; occorre una nuova legge speciale per la ricostruzione all'Aquila e nel e nel cratere. L'esasperazione che i cittadini hanno mostrato nella recente manifestazione è ampiamente giustificata. Noi ci impegneremo, e speriamo di poter incrociare la comune condivisione da parte della maggioranza, per fare in modo che questi argomenti vengano affrontati e definitivamente risolti. Concludo, signor Presidente, dicendo che vi sono molti motivi per dire no a questa manovra, per dire no alla fiducia al Governo. Questi motivi durante il corso dell'esame del provvedimento, nonostante il lavoro enorme compiuto in Commissione, si sono vieppiù accresciuti.

che risultava, nel dibattito avvenuto in Commissione, avere problemi di copertura finanziaria. rispetto a quel che si è detto, l'insieme dei precedenti conferma che, di fronte al Governo che insiste nella sua richiesta di fiducia sul complesso dell'emendamento portato alla Presidenza del Senato,

di farlo poi nelle sedi opportune. Ma voglio dire di più: alla luce del Regolamento attuale, non può che essere così. Naturalmente ben so, per esserne stato il proponente e averne discusso, che si possono realizzare modifiche regolamentari e, quando dovessero esserci,

Credo che questo fosse il punto in discussione. Vi è poi una cosa in più, signor Presidente: in realtà, il Governo ha anche fornito delle giustificazioni di natura tecnico‑finanziaria che, a suo modo di vedere, superano le osservazioni che erano state fatte. Voglio dire che non a caso il nostro

un'osservazione fatta qui in Aula, che pur aveva la sua fondatezza in relazione alla discussione del Senato, non poteva discussione del Senato, non poteva che ascoltare, oltre alla mia relazione che si limitava a riportare il dibattito,

ha la disponibilità dell'emendamento su cui pone la fiducia: con il nostro attuale Regolamento ne ha la totale disponibilità. Quindi, io credo che, sulla base di questo, oggi si sia operato correttamente. correttamente. Correttamente la Presidenza ha preso atto sia della discussione avvenuta in Commissione sia della volontà del Governo e pertanto si è proceduto sul testo presentato con la Quando il Regolamento cambierà, ove dovesse cambiare nel senso, per esempio, previsto anche nell'altro ramo del Parlamento, (dove il testo su cui viene

Stante la notevole rilevanza del problema che lei adesso ha affrontato e commentato, e che era stato

si può accettare il principio in base al quale, una volta che il Governo abbia posto la questione di fiducia, depositato il testo e dichiarato l'esistenza della copertura finanziaria,

Ripeto, il problema c'è, e questo, signor Presidente, lo comprenderebbe chiunque: se una somma sequestrata, che per definizione deve rimanere a disposizione del soggetto sottoposto ad indagine, viene

il problema si pone nel merito e sotto il profilo dell'applicazione del nostro Regolamento.